di introdurre questa relazione sull'amministrazione della giustizia, richiamando una lettera tra le numerosissime indirizzate al Ministro della giustizia. Era l'8 marzo scorso ed ero da poco insediata: «Illustre signora Ministro, le scrivo questa lettera pubblica per chiedere il Suo conforto, affranta dalla morte sul lavoro di mio figlio Roberto» (avvenuta quattro anni prima) «e dall'impossibilità di vedere celebrato il processo in tempi ragionevoli. anni e sono vedova. Roberto, il più piccolo dei miei figli, era il mio sostegno in tutto, aveva trentadue anni e viveva con me. Il nostro processo (…) non si riesce a celebrare, nonostante rientri in quelli cosiddetti a trattazione prioritaria (…). Il Tribunale (…) non è in grado (…) di poter far svolgere in sicurezza i processi con più parti a causa della carenza di aule attrezzate, risorse e personale e per questa ragione in un anno e mezzo, da quando è iniziato il dibattimento, a causa di continui rinvii è stato sentito solo uno dei circa venti testimoni. Con questa cadenza il processo di primo grado durerà numerosi anni Sono sicura che morirò prima di vedere la fine di questo processo (…) senza poter sapere come e da chi è stato ucciso mio figlio Le scrivo come madre, vedova e umile cittadina, per chiedere il Suo conforto e, nei limiti delle Sue possibilità e competenze, di approfondire la disastrosa realtà di quel tribunale. Prima di morire, vorrei poter andare sulla tomba di mio figlio Roberto per dirgli che la giustizia terrena ha fatto il suo corso».

È per ciascuno di loro che l'azione del Ministero della giustizia è stata orientata con determinazione verso un obiettivo che ho ritenuto cruciale: riportare i tempi della giustizia entro limiti di ragionevolezza. Come chiede la Costituzione; come chiedono i principi europei: il principio della ragionevole durata del processo e gli altri principi costituzionali ed europei che presidiano la corretta amministrazione della giustizia sono scritti per questo - per rispondere all'esigenza di chi, come questa anziana madre, attende dai nostri uffici giudiziari "una parola di giustizia" "una parola di giustizia" (P. Ricoeur). Processi irragionevolmente lunghi rappresentano un *vulnus* per tutti: per gli indagati e per gli imputati, che subiscono oltre il necessario la «pena del processo» e il connesso effetto di stigmatizzazione sociale; per i condannati, che si trovano a dover eseguire una pena a distanza di tempo, quando ben possono essere - e per lo più sono - persone diverse da quelle che hanno commesso il reato; per gli innocenti, che hanno ingiustamente subito oltre misura il peso di un processo che può aver distrutto relazioni personali e professionali; e soprattutto per le vittime e per la società, che non ottengono in tempi ragionevoli un accertamento di fatti ed eventuali responsabilità, com'è doveroso in un sistema di giustizia che aspiri ad assicurare la necessaria coesione sociale. La lettera di quell'anziana madre ci indica dove in molti casi si annidano i problemi che ostacolano il lavoro di magistrati e avvocati.

e questo fa riflettere. I grandi, nobili principi costituzionali ed europei (la durata del processo, il diritto di difesa, l'accesso alla giustizia) hanno bisogno di solido realismo e di pragmatica concretezza per non ridursi a vuota retorica. Come sarebbe stato il maxiprocesso di Palermo senza quell'aula *bunker* che fu oggetto dell'impegno dell'allora ministro della giustizia Mino Martinazzoli? I grandi principi hanno bisogno di organizzazione e risorse; hanno bisogno di magistrati, uomini e donne nelle cancellerie, oltre che nelle aule di udienza; hanno bisogno di strumenti informatici funzionanti e di edifici agibili. Sembrano cose scontate, ma non lo sono nello stato attuale del nostro sistema giustizia. giustizia. Questo è principalmente lo sforzo che il Ministero sta compiendo, in linea di continuità con il precedente Governo, che aveva predisposto un piano straordinario per le assunzioni. Spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi per la giustizia, come recita l'articolo 110 della Costituzione; è compito del Ministro, quindi, è servizio alla funzione del giudicare, servizio a tutti i suoi attori, procuratori, giudici e avvocati, e soprattutto è servizio ai cittadini. L'anno della giustizia 2021 è stato segnato da due fattori di contesto che hanno dominato tutto il sistema Paese: la pandemia e la pianificazione del PNRR con la sua prima attuazione, due elementi che, da un lato, hanno posto continui imprevisti, sfide e problemi, ma dall'altro hanno anche offerto una serie di opportunità e di spinte al cambiamento. Le emergenze si sono susseguite senza interruzione e quest'ultima ondata di contagi ha acuito ulteriormente le criticità, ma ogni giorno abbiamo cercato nuovi rimedi ai sempre nuovi problemi, abbiamo ricominciato e incessantemente reinventato il nostro modo di lavorare. Mi sia consentito di cogliere questa occasione per ringraziare pubblicamente e sentitamente i magistrati, gli avvocati, il personale amministrativo, la Polizia penitenziaria, tutto il personale degli istituti penitenziari e i volontari, che hanno continuato a far funzionare la macchina della giustizia e dell'esecuzione penale con spirito di adattamento e senza sottrarsi a rischi non trascurabili. Anche per la continuità di altre fondamentali attività ordinarie sono serviti impegno, creatività e capacità di riorganizzazione. Era indispensabile rimettere in moto le prove per l'esame per l'avvocatura, i concorsi per la magistratura (uno per 310 posti si è svolto la scorsa estate e un secondo per altri 500 è stato bandito da poco) e poi i concorsi per l'ingresso di altro personale (sono in corso le prove orali per 2.242 funzionari che erano state sospese per Covid). Inoltre, occorreva reinventare le modalità per i colloqui, le visite e le varie attività lavorative, culturali ed educative in carcere, per citare solo alcune delle emergenze recenti. Mentre l'emergenza sanitaria premeva con tutte le sue imperiose criticità, però, abbiamo messo a punto progetti e riforme strutturali a lungo termine, connessi agli obiettivi e alle opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da avviare il nostro sistema giustizia verso le grandi linee di modernizzazione concordate con le istituzioni europee. L'abbiamo detto mille volte: l'obiettivo, nell'arco di cinque anni, è l'abbattimento del 40 per cento del tempo medio di durata dei processi civili e del 25 per cento di quello dei processi penali. Ad oggi possiamo dire senza dubbio di aver conseguito - invero, anche in parte superato - gli impegni e gli obiettivi previsti per il 31 dicembre 2021. Il PNRR chiedeva l'approvazione delle leggi delega in materia di processo civile e processo penale, interventi in tema di insolvenza e l'avvio del reclutamento del processo, e lo abbiamo fatto. Uno sguardo di insieme a quest'anno intenso di lavoro, ricco di impegni e di traguardi, può essere riassunto secondo tre chiavi di lettura. La prima potrebbe essere definita così: dalla crisi un'opportunità, ovvero dalle misure emergenziali possibilità di riforme strutturali. Infatti, un indirizzo di quest'amministrazione è stato quello di cogliere le opportunità di rinnovamento del sistema giustizia emerse nella situazione della crisi in cui la pandemia ci ha posto, valutando quali misure, anche tra quelle imposte dalla contingenza, potranno tradursi in modifiche strutturali. Si pensi alle modalità di accesso alla professione di avvocato, che sono state cambiate, ma anche alle nuove modalità di svolgimento delle udienze, sia civili sia penali, e più in generale all'accelerazione della transizione digitale nei palazzi di giustizia e negli istituti penitenziari. Valuteremo quali di questi aspetti hanno funzionato e potranno essere mantenuti. In questa prospettiva, del resto, il PNRR chiede all'Italia - per il sistema giustizia - non interventi tampone, destinati a esaurirsi nell'orizzonte temporale del Piano, ma uno sforzo preordinato per un miglioramento definitivo. Credo che, con l'occasione della riflessione sul PNRR, si sia finalmente compreso che il sistema giustizia è un'infrastruttura portante dell'intero sistema Paese. Del resto, sappiamo bene che la modernizzazione e l'efficienza del sistema giudiziario incidono direttamente sulla solidità economica del Paese. Tra i tanti studi, ne cito uno della Banca d'Italia, che stima che la riduzione della durata dei processi di circa cento porta di per sé un incremento di almeno mezzo punto percentuale del PIL, e i nostri obiettivi di riduzione superano di gran lunga quel 15 Dunque, anche questa è la posta in gioco. La seconda chiave di lettura è il fattore Europa. L'anno della giustizia è stato dominato da un orizzonte europeo, e non soltanto per tutte le attività connesse all'attuazione del PNRR; ci sono molte altre iniziative che l'Unione europea sta promuovendo nel settore della giustizia. Ne cito alcune: prosecutor's office, EPPO), che ha iniziato ad operare nel corso di quest'anno, costituisce uno strumento fondamentale per il contrasto ai reati finanziari, alle frodi fiscali (un problema enorme), alla corruzione e all'uso illecito di finanziamenti europei, molto spesso oggetto di interessi delle mafie e della criminalità organizzata di varia natura. Nei primi sette mesi di funzionamento di EPPO, gli uffici italiani hanno avviato il più alto numero di indagini rispetto agli altri Paesi,

Come ho già avuto occasione di osservare, la Procura europea rappresenta una innovazione lungimirante e necessaria, nel momento in cui ingenti quantità di fondi europei stanno per essere messi in circolazione. Ce lo ha insegnato tanto tempo fa Giovanni Falcone, il primo a comprendere, già nel lontano 1991, in sede europea, la necessità di proteggere gli interessi finanziari dell'Europa con apposite strutture e misure. L'istituzione della Procura europea, con i suoi 22 procuratori delegati in Italia, davvero ha le sue origini più remote in una profetica intuizione del grande magistrato italiano, il cui sacrificio continua a dare frutti a trent'anni dalla strage di Capaci, che ricorderemo a maggio, seguita a luglio da quella di via D'Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino.

Sempre di matrice europea sono altri importanti interventi normativi approvati per dare attuazione ad impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea: ad esempio, la normativa in materia di lotta al riciclaggio, la normativa sulla presunzione di innocenza e quella relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Dobbiamo invece ancora dare attuazione alla direttiva sul *whistleblowing*, e bisognerà farlo al più presto, che rappresenta un prezioso strumento di contrasto alla corruzione, anche se una normativa è già in parte presente nel nostro sistema, in virtù di interventi varati nel 2012 e nel 2017. Siamo inoltre intervenuti sulla disciplina dell'acquisizione dei tabulati telefonici a fini di indagine, per adeguarci alle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tra le importanti iniziative prese sulla scia di stimoli variamente provenienti dall'Europa, dobbiamo anche ricordare quella sulla magistratura onoraria, che attendeva una risposta da troppo tempo. Grazie alla disponibilità del Governo che ha reperito le risorse necessarie, e di tutte le forze politiche in Parlamento, con la legge di bilancio siamo riusciti ad avviare una stabilizzazione per migliaia di magistrati onorari, che per anni hanno prestato il loro essenziale servizio in una condizione di totale assenza di tutele lavorative (né malattia, né maternità, né ferie), una carenza più volte stigmatizzata dalle Istituzioni europee. La terza chiave di lettura che riassume l'attività di questi mesi è, come avrete già intuito, la centralità del fattore organizzativo. La riduzione dei tempi del processo richiede riforme, ma soprattutto una nuova organizzazione. Come ben sapete, la giustizia è stata interessata da alcune importanti riforme che il Parlamento ha approvato superando le non irrilevanti divergenze di vedute e di sensibilità tra le varie forze politiche, lasciando prevalere un senso di responsabilità verso il bene comune e il primario interesse del Paese. Ciò che però mi preme sottolineare è che quelle riforme per diventare effettive richiedono un'imponente ristrutturazione dell'organizzazione del servizio giustizia, accompagnata dall'immissione di ingenti risorse umane e materiali. Organizzazione e capitale umano sono la condizione di effettività di quelle riforme. Per questo, prima di ripercorrere brevemente i principali capitoli delle riforme normative approvate nel corso di quest'anno, vorrei attirare la vostra attenzione sulla riorganizzazione del settore giustizia attualmente in corso. Il primo e più importante cambiamento è stata l'istituzione dell'ufficio del processo. Questa è l'innovazione più rilevante, il pivot della nuova organizzazione della giustizia, che a brevissimo porterà nei nostri uffici giudiziari migliaia di giovani giuristi in ausilio al lavoro dei magistrati. Il sistema italiano già conosceva questa struttura, perché l'abbiamo sperimentata in vari distretti di corti d'appello; ora però la diffondiamo gradualmente in tutti gli uffici e questo comporterà un vero e proprio cambio di paradigma nell'organizzazione del lavoro, perché segna il passaggio dal lavoro individuale e solitario del giudice a quello di squadra. Più volte in questi mesi, nel dibattito pubblico, si sono sentite voci preoccupate per l'incalzare di una sorta di visione efficientistica della giustizia. Mi preme rimarcare che, se ben organizzato e ben condotto, l'ufficio del processo non solo incrementa l'efficienza della giustizia, migliorandone i tempi (che, come abbiamo visto, non sono fattori secondari), ma ne favorisce anche la qualità. E non c'è competizione, né tantomeno contraddizione, tra efficienza e qualità della giustizia, ma reciproco sostegno, nel quadro dell'ufficio del processo. processo. A brevissimo, il 14 febbraio, 200 giovani giuristi entreranno in Cassazione; il 21 febbraio, altri circa 8.000 prenderanno servizio in tutti gli uffici giudiziari italiani. Notate le cifre: in servizio oggi abbiamo circa 9.000 magistrati e l'ingresso di circa 8.200 giovani giuristi assistenti è un aiuto potenzialmente molto rilevante, sia quantitativamente, sia - non mi stanco di ripeterlo - per il collegamento intergenerazionale che questo ufficio può portare. Sempre nel medesimo quadro dell'ufficio del processo, nelle prossime settimane ci sarà un contingente di tecnici importante (5.410) che supporterà questo ufficio in compiti come *data entry*, rilevazione statistica e analisi organizzativa (tutti i compiti di supporto dell'azione gestionale dei vertici giudiziari e amministrativi degli uffici). Non posso non ringraziare qui il Dipartimento della funzione pubblica per averci sostenuto nella celebrazione di questi concorsi, che hanno visto la partecipazione di decine e decine di migliaia di aspiranti. Ovviamente però i numeri non bastano: occorre che le persone siano formate e ben organizzate, e così stiamo lavorando con la Scuola superiore della magistratura e la Scuola nazionale dell'amministrazione, che pure ringrazio per la collaborazione, per offrire un'adeguata formazione non solo al personale selezionato (questi giovani giuristi), ma anche ai vertici degli uffici giudiziari, che sono chiamati a un enorme sforzo di riprogettazione del loro modo di lavorare e delle loro strutture, per poter destinare proficuamente le nuove risorse umane ai bisogni specifici di ogni tribunale, di ogni sezione e di ogni corte. Questo ufficio sarà stabilizzato nel tempo, come prevedono già le riforme del processo penale e civile, che hanno anche contingenti muniti di copertura finanziaria; l'idea è che questa grande innovazione sia destinata a cambiare il volto dei nostri uffici giudiziari anche oltre l'orizzonte del PNRR. La seconda misura organizzativa importante

Permettetemi di soffermarmi soltanto un istante sulla centralità e l'importanza che, anche nell'ambito della giustizia, si sviluppi una corretta cultura del dato, della statistica e della sua trasparenza, che è condizione fondamentale per il buon andamento di tutti i servizi pubblici, inclusi quelli della giustizia. Lo sappiamo, gli obiettivi della riduzione dei tempi dei processi non si conseguiranno d'un tratto; non è opera che si può compiere da un giorno all'altro: ne siamo tutti consapevoli. altrettanto consapevoli di aver posto le basi e avviato un processo virtuoso, ma sappiamo che il suo completamento richiederà tempo. Sarà un cammino graduale, che, per non deragliare, dovrà essere accompagnato da una costante rilevazione dell'andamento dei tempi di ciascun ufficio giudiziario, in modo da poter intervenire tempestivamente per rispondere con risorse più adeguate alle esigenze emergenti, per rimuovere ostacoli imprevisti e per affrontare tanti problemi, che - realisticamente - non mancheranno. Per questo è indispensabile anche nel settore giustizia sviluppare politiche pubbliche fondate sul dato e sulla trasparenza, costantemente verificate sulla base dell'esperienza statisticamente elaborata. Abbiamo imparato in questi mesi che garantire una misurazione accurata dell'impatto delle riforme è imprescindibile per la fiducia delle istituzioni europee nel nostro Paese, ma ai miei occhi è di più: è anche un dovere di trasparenza verso i cittadini, un impegno di democrazia che nel tempo rinsalda la fiducia reciproca tra istituzioni e cittadinanza. La fiducia è un bene di cui c'è un immenso bisogno. Permettetemi di ricordare un piccolo episodio che mi è capitato in un dialogo in un contesto di imprenditori e investitori internazionali. A un certo punto, in questo dialogo in cui stavo illustrando le riforme della giustizia in Italia, gli obiettivi e i mezzi che abbiamo messo a disposizione, mi è stata posta questa domanda: «Ma quando potremo tornare a investire in Italia, certi che i tempi della giustizia saranno davvero comparabili a quelli degli altri Paesi? Quando?». Questa domanda dice quanta attenzione c'è anche da parte degli osservatori internazionali, com'è emerso anche in alcuni giornali, che invitano gli investitori tornare a volgere lo sguardo all'Italia. Cosa rispondere a una domanda simile? Possiamo offrire risposte evasive, generiche o ingannevoli? Domani, fra un anno, fra sei mesi o fra due anni? Non mi sono sentita di dare un tempo, ma di dire che l'unica risposta credibile è: il tempo lo deciderete voi; noi vi assicureremo di avere a disposizione i dati, le statistiche, tutti gli elementi in piena trasparenza, perché possiate fare le vostre valutazioni e e assumere le vostre decisioni. Questa è l'amministrazione della giustizia che ho in mente e l'istituzione del nuovo dipartimento presso il Ministero contribuirà a sviluppare questa cultura del dato, con la possibilità di accedere direttamente alle stime di tutti i servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche a quelli raccolti dagli uffici con il dovere di renderli accessibili, ovviamente nel pieno rispetto dei principi e delle esigenze della riservatezza delle indagini e dei dati personali. Il monitoraggio sui dati è particolarmente indispensabile nell'ambito della riforma penale e per questo la legge delega prevede un apposito comitato tecnico-scientifico, che abbiamo già insediato a dicembre, per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, con il compito di effettuare una verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione, nel rispetto dei principi del giusto processo. Questo comitato di monitoraggio ha al suo interno una unità dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione. Da parte nostra e delle istituzioni europee c'è una costante preoccupazione sulla piaga della corruzione, che richiede attenzione, per la sua capacità - come aveva detto tempo fa il Presidente della Repubblica - di divorare risorse pubbliche e minare il rapporto di fiducia tra Stato e cittadini. Ufficio del processo, cultura del dato e monitoraggi. Il terzo aspetto è quello della digitalizzazione l'istituzione del nuovo Dipartimento rispecchia anche questa attenzione costante alla digitalizzazione, che nell'ambito della giustizia non implica soltanto la dematerializzazione degli atti cartacei in tutti i procedimenti civili e penali, ma consente un nuovo sistema di organizzazione delle forme processuali e potenzia gli strumenti di conoscenza a disposizione delle procure e dei giudici. La qualità della digitalizzazione, eventualmente anche coadiuvata dall'intelligenza artificiale nel rispetto della carta etica adottata dalla Commissione condiziona già oggi e condizionerà sempre più la qualità della risposta dei servizi della giustizia e la sua tempestività. Ci sono molti progetti in corso e ne richiamo soltanto due, che sembrano piccoli, ma vanno a snidare alcuni problemi molto particolari del nostro sistema. Uno è il recentissimo avvio del nuovo applicativo SIAMM Pinto digitale, che è una piattaforma per la gestione delle procedure di pagamento degli indennizzi dovuti alla violazione della ragionevole durata del processo. Si tratta di procedure che, a loro volta, spesso avevano lo stesso vizio del male che volevano sanare, vale a dire generavano ulteriori irragionevoli durate del processo. Poi, nel quadro della spinta alla digitalizzazione del processo penale, vorrei citare un progetto volto ad abbattere e a risolvere il problema dei cosiddetti tempi del carrello, quei tempi, che a volte sono lunghissimi e si misurano in termini di mesi, se non di anni, per il transito del procedimento da un grado all'altro del giudizio. Sembra un aspetto di poco conto, ma tante volte la durata del giudizio di appello, che è il nodo più difficile e meno virtuoso del nostro processo penale, non è dovuta alla durata delle udienze o al lavoro del giudice, ma ai tempi del passaggio delle carte. Pertanto, con la DG Reform della Commissione europea abbiamo elaborato un progetto, che mira ad azzerare questo problema dei tempi di attraversamento del fascicolo e credo che potrà dare un grande beneficio proprio ai giudizi di appello, su cui si appuntano tante criticità del nostro sistema. Sono due piccoli esempi, tra i tanti che potrei menzionare, ma non lo farò perché abbiamo tante altre cose da dirci. Vorrei però sottolineare che lo sviluppo dei nuovi progetti che il Ministero della giustizia sta promuovendo anche con la collaborazione del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale deve accompagnarsi e svilupparsi parallelamente a interventi indifferibili per la risoluzione dei problemi informatici quotidiani, dovuti - come sanno bene gli avvocati, presenti anche in quest'Aula - alla obsolescenza e alla frammentazione di quelli già in essere. I sistemi in atto hanno bisogno di manutenzione continua e di un ripensamento radicale. Permettetemi di concludere questa parte, che è la più corposa, su tutti gli aspetti organizzativi, con una notazione di metodo. Sin dall'inizio del mio mandato ho cercato di assicurare che il Ministero della giustizia operasse sempre in sinergia con tutti gli attori del sistema giustizia: Consiglio superiore della magistratura, Scuola superiore della magistratura, singoli uffici giudiziari, Avvocatura e anche con l'università. La collaborazione istituzionale, che è un principio costituzionale e una buona regola da seguire per il regolare funzionamento di ogni ramo dell'amministrazione, per la giustizia è una esigenza imperativa, in considerazione del fatto che l'indipendenza e l'autonomia del potere giudiziario dei singoli magistrati accentuano la necessità del coinvolgimento e del coordinamento fra tutti i protagonisti. Per questo, nei mesi scorsi, ho iniziato a visitare una a una personalmente tutte le Corti d'appello, per conoscere, vedere e discutere col territorio le indicazioni, i principali problemi e le principali criticità. Nella stessa prospettiva, un ruolo fondamentale è stato svolto

Ancora, mi preme segnalare un importante protocollo, firmato da CSM, Scuola della magistratura e Ministero, per la formazione dei dirigenti degli uffici giudiziari. Una relazione virtuosa si sta sviluppando anche con l'università. A titolo esemplificativo ricordo il finanziamento per 51 milioni di euro di sei macro progetti, che coinvolgono 57 atenei statali, per la diffusione dell'ufficio del processo, per l'implementazione dei modelli operativi innovativi negli uffici giudiziari e per lo smaltimento dell'arretrato. Passo ora a ricordare - davvero velocemente, perché le conoscete meglio di me - le riforme normative che il Parlamento ha approvato negli scorsi mesi. So bene quanta fatica e quanta disponibilità siano state chieste a tutte le forze politiche per trovare un terreno su cui convergere. Queste riforme sono figlie del contesto straordinario in cui sono nate: un Governo sostenuto da una maggioranza amplissima, di unità nazionale, con sensibilità al suo interno molto distanti fra loro. Ma il cammino delle riforme della giustizia - un cammino non sempre lineare, lo sappiamo - è stato sorretto dalla comune responsabilità per l'interesse del Paese, alla ricerca sempre di un'equilibrata sintesi, e di questo ringrazio sentitamente tutte le forze politiche. Quanto ai singoli capitoli delle riforme, davvero mi limito a enunciarne i titoli e il significato essenziale. La prima e più importante è la riforma del processo penale, approvata in Parlamento con l'obiettivo di coniugare maggiore efficienza del sistema con il rispetto delle fondamentali garanzie costituzionali in materia penale. L'impianto poggia su due pilastri: da un lato incide sulle norme del processo penale, operando sulle sue varie fasi, dalle indagini fino al giudizio in Cassazione, allo scopo di sbloccare possibili momenti di stasi, incentivare i riti alternativi, far arrivare a processo solo i casi meritevoli dell'attenzione del giudice; dall'altro la riforma prevede interventi sul sistema sanzionatorio penale, capaci di produrre anche significativi effetti di deflazione processuale. Questa parte della riforma prosegue lungo una linea già presente nel nostro ordinamento, volta a radicare l'idea, costituzionalmente orientata, che la certezza della pena non è la certezza del carcere: l'articolo 27 della Costituzione parla di pena e non di carcere. È in questa prospettiva che va, quindi, letta la valorizzazione delle pene alternative alla reclusione che ormai, come ampiamente dimostrato, portano in alcuni casi, laddove possibile, a una drastica riduzione della recidiva. Ne beneficiano i singoli e ne beneficia la società. Peraltro, come ben sapete, la riforma della giustizia penale ha affrontato anche il nodo della prescrizione. Da un lato, è stato confermato il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado previsto con la riforma del 2019 e, dall'altro, sono stati apportati alcuni correttivi a garanzia dell'imputato, introducendo nei giudizi di impugnazione il nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi. L'istituto dell'improcedibilità è stato modulato in modo da assicurare sempre che tutti i processi arrivino a sentenza definitiva. Il monitoraggio statistico di cui abbiamo parlato aiuterà ad assicurare che questo obiettivo sia sempre conseguito. In materia penale, tra le riforme ancora da attuare non possiamo non menzionare almeno quella sull'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, di prossima discussione in Commissione giustizia alla Camera. A maggio scadranno infatti i dodici mesi di tempo dati dalla Corte costituzionale al Parlamento per intervenire sulla materia, nel rispetto dei principi costituzionali e salvaguardando le specificità e le esigenze del contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata in generale. Non posso concludere questa parte sulla giustizia penale senza fare un cenno al fatto che uno dei fili rossi che legano le trame della riforma è la è la riparazione dell'offesa e l'attenzione alle vittime. Si spiega così il capitolo della riforma che reputo più innovativo, quello dedicato alla giustizia riparativa, sul quale tornerò brevemente in conclusione. Anche la riforma del processo civile, la seconda grande riforma, punta a fornire risposte più celeri alle esigenze quotidiane dei cittadini e delle imprese, intervenendo su un doppio binario: da un lato, valorizzando e perfezionando gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) al fine di deflazionare il carico dei tribunali e favorendo soluzioni consensuali dei conflitti; dall'altro, agisce sulle procedure con interventi mirati e circoscritti nell'ottica della semplificazione. La riforma mira a realizzare una maggiore concentrazione delle attività processuali nell'ambito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa: riduzione della domanda, razionalizzazione della risposta. Tra le innovazioni della riforma segnalo soltanto la grande novità del rinvio pregiudiziale in Cassazione, che permette di coinvolgere precocemente la Corte di cassazione quando sorgono dubbi interpretativi, senza aspettare la fine dei tre gradi di giudizio, di modo che il giudice possa prevenire la formazione di contrastanti orientamenti territoriali e favorire la certezza del diritto con un importante effetto deflattivo. terzo capitolo riguarda la riforma dell'insolvenza dovuta e necessitata dalla situazione di crisi economica che si è sviluppata con la pandemia. È un intervento normativo indispensabile e l'obiettivo è quello di offrire nuovi e più efficaci strumenti agli imprenditori per sanare quelle situazioni di squilibrio economico e patrimoniale che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili. Il cuore di questa riforma è la composizione negoziata della crisi, un percorso volontario attraverso il quale l'imprenditore, lontano dalle aule giudiziarie e in assoluta riservatezza, si rivolge a un esperto terzo e imparziale. Questo istituto è accompagnato da sistemi di allerta, sia interni che esterni alle aziende demandati dai creditori pubblici qualificati, affinché l'imprenditore possa fare un'autodiagnosi e avvalersi per tempo di questo strumento. La tempestività è il cuore della riuscita di queste operazioni. Un capitolo della riforma del processo civile è stato dedicato alla famiglia e ai minori: troppi i casi di violenza sulle donne, troppi i femminicidi, troppe le violenze sui bambini, troppi i drammi che originano in un ambito domestico e di cui abbiamo notizia quotidianamente. Una vera barbarie, ha detto qualcuno di voi. Il contenzioso nell'ambito delle relazioni familiari sta crescendo e si fa sempre più complesso: cause di separazione si intrecciano a denunce di violenza domestica, specialmente nei confronti delle donne, o ad azioni del giudice a protezione dei minori. Troppo spesso un insufficiente coordinamento di tutte le autorità procedenti - tribunale per i minorenni, tribunale ordinario civile, giudice penale, giudice tutelare - rende inefficace l'intervento di tutti e riduce la possibilità di di prevenire conseguenze anche fatali. Di qui l'esigenza di una profonda riforma delle procedure e dell'organizzazione giudiziaria del settore, che sfocerà a tempo debito nell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, allo scopo di incrementare le garanzie processuali dei soggetti più vulnerabili facendo tesoro della grande esperienza dei giudici minorili e valorizzandone ancor di più la specializzazione in un nuovo e più razionale contesto ordinamentale. Delega penale, delega civile, diritto di famiglia dei minorenni, insolvenza: sul piano delle riforme abbiamo veramente fatto moltissimo. Le più importanti di queste riforme sono state assunte nella forma della legge delega e quindi oggi richiedono l'attuazione dei decreti legislativi delegati che per il PNRR devono essere pronti entro la fine del 2022. Posso assicurarvi che su questo stiamo già lavorando con diversi gruppi di lavoro sia nel penale che nel civile e spero di poter anticipare i tempi, ma sappiamo bene che all'appello manca un altro fondamentale - e da tutti atteso - capitolo delle riforme, la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, che il Presidente della Repubblica e alcune forze politiche ancora di recente giustamente Il disegno di legge delega è già incardinato alla Camera, su iniziativa del precedente Governo, e come abbiamo fatto con le altre riforme intendiamo presentare emendamenti governativi. Voi lo sapete: nel corso dell'autunno, dopo l'approvazione della delega penale e civile, subito abbiamo creato occasioni di confronto con i responsabili per la giustizia delle varie forze politiche abbiamo avuto più interlocuzioni con l'Associazione nazionale magistrati, con il Consiglio superiore della magistratura e con l'Avvocatura per addivenire a proposte di emendamenti da presentare alla Camera. Queste proposte sono oggi all'attenzione del Governo. Gli emendamenti intervengono su vari aspetti del disegno di legge e riguardano, tra l'altro, il sistema elettorale, la composizione e il funzionamento del CSM, il conferimento degli incarichi direttivi, le valutazioni di professionalità, il collocamento fuori ruolo dei magistrati, il concorso per l'accesso in magistratura, il rapporto tra il magistrato e le cariche elettive. Sono certa che nelle prossime settimane potremo progredire nella scrittura anche di questo atteso capitolo della riforma, che peraltro anche il PNRR ci chiede di approvare quest'anno. La Camera ha già calendarizzato la discussione in Aula e quella scadenza dovrà essere rispettata. Per parte mia, come ho sempre fatto, continuerò voi lo sapete bene, perché con voi ho tante volte interloquito su questi temi - non solo a dare la mia massima disponibilità, ma anche a spendere tutte le mie energie per accelerare il corso di questa riforma e sollecitarne l'esame da parte dei competenti organi del Governo.

Uno è il capitolo penitenziario e l'altro è quello delle attività internazionali. Quanto al carcere, come ho già avuto modo di osservare, la pandemia ha fatto da detonatore a questioni irrisolte da lunghissimo tempo. Questi anni sono stati durissimi. Tensioni, paure, incertezze, isolamento che tutti abbiamo sperimentato, erano e sono amplificati dentro le mura del carcere, per tutti: per chi lavora in carcere e per chi in carcere sconta la sua pena. Se vogliamo farci carico davvero dei mali del carcere, in primo luogo perché non si ripetano mai più episodi di violenza come quelli che abbiamo visto quest'anno, ma, più ampiamente, perché la pena possa davvero conseguire la finalità prevista dalla Costituzione, occorre concepire e realizzare una strategia che operi su più livelli: investimenti sulle strutture penitenziarie, accelerazioni delle assunzioni del personale, più ricca formazione del personale in servizio, diffusione dell'uso delle tecnologie, tanto per le esigenze della sicurezza quanto per quelle del trattamento dei detenuti. Il primo e più grave di tutti i problemi continua a essere il sovraffollamento. Ogni tanto ce ne dimentichiamo ma oggi, su 50.832 posti regolamentari, di cui, invero, sono 47.418 quelli effettivi, i detenuti sono 54.329, vale a dire una percentuale di sovraffollamento del 114 Il sovraffollamento è una condizione esasperante, tanto per i detenuti quanto per la polizia penitenziaria, troppo spesso vittima di aggressioni. Sovraffollamento significa maggiore difficoltà a garantire la sicurezza e significa maggiore fatica a proporre attività che consentano alla pena di favorire percorsi di recupero. Occorrono più spazi, occorre sviluppare pene diverse dalla reclusione in carcere. Come ho già detto, la riforma approvata va in questa direzione, ma la realtà delle forme alternative al carcere è già presente in modo significativo nel nostro ordinamento. Vorrei sottolineare in questa sede che le persone in esecuzione penale esterna superano il numero dei detenuti. Sono oltre 69.000, a fronte di circa 54.000 detenuti. E negli UEPE, gli uffici per l'esecuzione penale esterna, sono solo 1211 le unità di personale che se ne occupano. È evidente la necessità di potenziare questo settore e le forze politiche hanno avuto la sensibilità di sottolinearlo, in un ordine del giorno approvato a margine della legge di bilancio. Naturalmente, occorre fare molto anche per le strutture edilizie: alcune davvero non sono degne del nostro Paese. Venerdì scorso ho visitato il carcere di Sollicciano a Firenze: è in condizioni indecorose, nonostante la ristrutturazione straordinaria in atto. E qui si verificano, non a caso, importanti numeri di autolesionismo e di suicidi. Bisogna ripensare gli spazi. Il tema degli spazi richiede, anzitutto, interventi finalizzati a garantire le essenziali condizioni di decoro ed igiene, ma implica anche un ripensamento dei luoghi, in modo che essi non siano solo contenitori di uomini, ma ambienti densi di proposte, di lavoro, di attività, di cultura. Solo così si assolve a pieno al valore costituzionale della pena. In questa prospettiva, mi piace ricordare il lavoro svolto dalla Commissione sull'architettura penitenziaria, che al mio arrivo al Ministero era già insediata e stava finendo i suoi lavori. Essa ci ha offerto fecondi suggerimenti, che stiamo cercando di attuare. Con i fondi complementari del PNRR stiamo realizzando otto nuovi padiglioni, ampliamenti degli istituti esistenti, che riguardano tanto i posti disponibili, le camere, quanto i posti trattamentali. Per questo aspetto abbiamo corretto i precedenti progetti. Da mesi mi sto dedicando anche al problema della salute mentale in carcere, insieme ai Ministri della salute e per gli affari regionali e agli altri attori istituzionali coinvolti. È un dramma davvero

È vero che il numero di persone in attesa di un posto nelle REMS è calato (erano 98 nell'ottobre 2020, oggi 35), è vero che abbiamo all'orizzonte - spero di poterlo annunciare nei prossimi giorni - la disponibilità di una nuova struttura che potrà dare sollievo anche a questa problematica, ma, credetemi, il lavoro da fare qui è ancora tantissimo.

Occorre investire di più nella formazione - nella relazione trovate tutti i dati e i numeri - soprattutto della polizia penitenziaria, come mi richiedono costantemente i sindacati. Il compito che svolge è delicatissimo, perché non è solo vigilanza, custodia e sicurezza: è presenza quotidiana accanto al detenuto. Questo personale deve essere sostenuto da un'adeguata e costante formazione. In questi mesi ho raccolto moltissime testimonianze che raccontano quanto sia stata decisiva la presenza di un agente per segnare una svolta nella vita di un detenuto. Ultimo passaggio sul carcere: lo scorso 17 dicembre la Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario che avevo istituito alcuni mesi fa ci ha proposto delle soluzioni per contribuire a migliorare la qualità della vita e dell'esecuzione penale nella sua quotidianità, con un *focus* particolare sulla gestione della sicurezza, l'impiego delle tecnologie, la tutela della salute, sul lavoro, sulla formazione professionale dei detenuti e sulla formazione del personale. Ci sono grandi potenzialità che possono dare sollievo a questo mondo, legate alle tecnologie (sorveglianza, *body cam*, sistemi anti droni, colloqui a distanza, lezioni e conferenze *on line*, tanto altro, telemedicina) e, grazie alla sensibilità e all'interessamento del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, si stanno progettando molti interventi che possono diventare altrettante occasioni di lavoro per i detenuti. L'ultimo capitolo è quello dell'attività internazionale, forse meno conosciuto - non si pensa a questa proiezione internazionale del Ministro della giustizia - e che invece è fondamentale sia per far crescere la cultura dei diritti fondamentali che per per coltivare una cooperazione giudiziaria rafforzata per il contrasto ai grandi fenomeni di criminalità transnazionale. Ci sono moltissimi progetti in atto, che vanno dai rapporti bilaterali - per esempio, con alcuni Paesi come l'Albania - per permettere ai detenuti, laddove ci siano le condizioni, di scontare la pena nel loro Paese d'origine. Ci sono casi sotto l'attenzione di tutti: di nuovo, in questi giorni, anche per la ricorrenza che stiamo per vivere a breve, il caso Regeni richiede al Ministero - come l'autorità giudiziaria ci ha sollecitato a fare di intensificare l'attività per permettere a questo processo di svolgersi. C'è stato il caso francese, in cui, dopo anni di attesa, gli organi politici francesi hanno rimosso gli ostacoli per permettere alle autorità giudiziarie francesi di esaminare l'*iter* di estradizione per le persone condannate in via definitiva per gravissimi reati commessi negli anni di piombo. Poi, c'è stato tutto il capitolo dell'Afghanistan che ha coinvolto anche il Ministero della giustizia per il legame ventennale che che il nostro Paese ha avuto con l'Afghanistan proprio per la costruzione dello Stato di diritto. Non potevamo e non volevamo dimenticarci di quei magistrati e avvocati che così tanto avevano collaborato con le autorità italiane durante la nostra presenza in Afghanistan. Ci siamo adoperati per fare avere la protezione internazionale a figure di particolare rilievo che erano a rischio con il nuovo regime. Tra queste l'ex procuratore generale della provincia di Herat, Maria Bashir, una figura di primo piano nella difesa dei diritti delle donne e nella costruzione di uno Stato di diritto nella sua terra, in collaborazione con il nostro Paese, cui poi il Presidente della Repubblica ha voluto concedere la cittadinanza italiana per altissimi meriti. Nel quadro delle tantissime iniziative internazionali, su cui non voglio intrattenervi oltre, ce n'è una che merita attenzione: è la Conferenza è la Conferenza dei ministri della giustizia dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, che abbiamo svolto a Venezia il 13 e 14 dicembre scorso, su criminalità e giustizia penale e sul ruolo della giustizia riparativa in Europa. Qui mi ricollego a quel capitolo della riforma penale a cui avevo fatto cenno. La Conferenza è stata il primo evento di livello ministeriale nell'ambito della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa: vi hanno preso parte il Segretario generale e 40 delegazioni. Questa importante iniziativa ha portato alla condivisione della Dichiarazione di Venezia sulla giustizia riparativa, che poi è stata adottata dai più alti organi del Consiglio d'Europa in questi giorni. Con questa Dichiarazione tutti gli Stati del Consiglio d'Europa si sono impegnati a sviluppare un nuovo paradigma della giustizia penale, complementare a quello tradizionale e che muove dall'esigenza di coinvolgere attivamente in percorsi guidati da mediatori professionisti il reo e la vittima, ma anche la comunità di riferimento, con l'obiettivo fondamentale di riparare e restaurare i legami sociali lacerati dal reato, di responsabilizzare l'autore dell'offesa, ma anche di porre le basi per una futura e più consapevole ripresa delle relazioni nei contesti di appartenenza. Le ricadute sono tangibili, ben chiare e ben documentate dagli studi empirici svolti a livello nazionale e internazionale: riduzione della recidiva, alleggerimento dei processi penali, nuova centralità per la vittima, lasciata troppo spesso sullo sfondo dei procedimenti giudiziari e sola con il suo dolore. dolore. Permettetemi allora di concludere proprio su questo capitolo della giustizia riparativa, che di certo è il più innovativo per il nostro sistema. La giustizia riparativa non è un atto di clemenza, né tantomeno esprime un pensiero debole in materia penale; al contrario, è uno strumento che si sviluppa a fianco delle tradizionali forme di contenimento della libertà del condannato, irrinunciabili quando sussistono esigenze di difesa sociale a fronte della pericolosità dell'autore del reato. La giustizia riparativa è una giustizia esigente, perché chiede al trasgressore di assumersi tutta la sua responsabilità di fronte alla vittima e di fronte alla comunità, attraverso incontri liberamente concordati, con l'aiuto di un terzo che favorisce il riconoscimento della verità dell'accaduto. Avrei un esempio carino da proporvi, ma vedo che il tempo è stato troppo lungo e lo lascio allo scritto per chi vorrà leggerlo: riguardava il caso di una cittadina nel Salernitano, dove era stato bruciato, in uno dei tanti incendi dolosi, il bosco vicino. Perché è così decisivo coltivare questo percorso della giustizia riparativa? Perché l'ordinamento, con questi strumenti, si apre alla possibilità di un sistema giudiziario in grado di domare la rabbia provocata dal reato e di ricostruire i legami civici tra i cittadini. Più in generale, si tratta di uno strumento che contribuisce a coltivare una cultura che può diventare un paradigma per prevenire e regolare i conflitti dell'intera *polis* sulla scorta di esperienze storiche straordinarie, come la Commissione per la verità e la riconciliazione di Nelson Mandela e di Desmond Tutu alla fine dell'*apartheid* in Africa. Noi abbiamo già molte sperimentazioni feconde di questi sistemi. Questa è la concezione della giustizia che mi sta a cuore e che ritroverete in filigrana in tutti gli interventi di riforma che ho qui in sintesi ripercorso. Una giustizia che ricuce e ripara, che non si nutre di odio che non cede alla reazione vendicativa, ma che vive innanzitutto di ricerca della verità, di quella verità che emerge nella narrazione di fronte all'altro, nell'incontro personale, nel racconto e nell'ascolto reciproco del proprio vissuto. Questa è la giustizia su cui sono stata chiamata a riflettere proprio sul luogo della massima ingiustizia della nostra storia, quel binario 21 alla stazione centrale di Milano da cui partivano i treni di Auschwitz. In una delle giornate più intense di tutto il mio servizio al Ministero sono stata invitata dalla senatrice a vita Liliana Segre e da lei accompagnata fino a quei vagoni da cui da bambina partì insieme al padre per una destinazione sconosciuta, ignota, il campo di concentramento. Quelle atrocità, di cui oggi tutto il mondo si vergogna e che tra qualche giorno ricorderemo nel Giorno internazionale della memoria, sono state alimentate, come si legge a chiare lettere davanti al binario 21, dalla indifferenza, dall'incapacità di ascoltarsi, dalle piccole e grandi discriminazioni, dai discorsi d'odio, dall'idea dell'altro come nemico. Coltivare un'idea della giustizia che abbia a cuore la ricerca della verità e abbia cura dei rapporti personali e sociali è quanto ho inteso perseguire in quest'anno quasi di servizio al Ministero della giustizia. Sono convinta che questa sia la più grande urgenza del nostro tempo e che questo è lo spirito che ci trasmette la nostra Costituzione. Grazie per la pazienza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la ministra, professoressa Marta Cartabia, per la puntuale relazione sull'amministrazione della giustizia. L'anno che si è appena concluso è stato segnato dalla pandemia per cui la risposta che il Parlamento e il Governo, d'intesa con tutti gli attori del sistema giustizia, hanno saputo offrire è risultata idonea al raggiungimento di importanti risultati, obiettivi prefissati già dall'inizio della legislatura. Se da un lato infatti si è inteso prorogare alcune delle misure emergenziali realizzate nell'anno precedente che hanno evitato la paralisi della giustizia, come quelle relative ai processi da remoto, che hanno consentito, seppur in condizioni non sempre ideali, la celebrazione dei processi, dall'altro si è provveduto ad una massiccia dose di assunzioni tramite l'espletamento di concorsi pubblici. La macchina della giustizia dunque non si è mai fermata; una riprova è nel fatto che più di 8.000 giovani giuristi inizieranno il loro percorso presso il neocostituito ufficio del processo proprio il mese prossimo. L'approvazione delle leggi di delega al penale e al civile segnano il primo importante passo verso un sistema più veloce e anche per molteplici aspetti, forse non tutti, più efficiente. Deve essere valorizzata la figura della magistratura onoraria che nel corso di questi anni ha svolto un'importante funzione. Il Parlamento è pronto a dare il suo contributo nella stesura dei decreti legislativi, auspicando una continua e proficua collaborazione con il legislatore delegato. La legislazione emergenziale si è dovuta adattare alle restrizioni imposte dal virus, modificando in radice anche importanti aspetti formativi dei ragazzi che si affacciano alla professione forense; emblema di ciò sono le modifiche alle modalità di accesso. Queste sono alcune delle norme che hanno caratterizzato l'intenso sforzo del legislatore al fine di mitigare le conseguenze dannose della pandemia. L'aspetto a cui tengo è quello relativo agli interventi in ambito penitenziario. *Despondere spem munus nostrum*, garantire la speranza è il nostro compito. Per più di vent'anni a capo di strutture complesse come quelle del carcere, ho fatto mio questo principio, scritto sullo stemma araldico del corpo della Polizia penitenziaria, con il quale quotidianamente ho avuto l'onore di interfacciarmi e lavorare. Il carcere è un luogo di comunità, dove la sofferenza di uno è la sofferenza di tutti, ma dove la speranza di ciascuno è la speranza di tutta la nostra società. Dall'inizio di questa legislatura ho impegnato tutte le mie energie al fine di contrastare i problemi atavici che permeano il nostro sistema carcerario. L'articolo 27 della Costituzione fa sì che il carcere non sia un luogo di repressione, ma di ordine, sicurezza e trattamento, dove i detenuti sono condotti all'interiorizzazione delle norme, alla responsabilizzazione e al rispetto delle regole mediante un processo di inclusione incentrato sull'autonomia, la socializzazione e l'integrazione. Lo scopo della pena è quello di eliminare la recidiva. In questo senso, anche la previsione di assunzione di assistenti sociali appartenenti al dipartimento di comunità espressione della necessità di assicurare la fattibilità delle misure alternative, anche nei confronti di coloro che non hanno domicili idonei. Infatti vi è un'oggettiva difficoltà nello smaltimento dei numeri del sovraffollamento carcerario, dato anche dal fatto che spesso l'accesso alle misure alternative richiede un domicilio idoneo presso il quale scontare la pena. Per cui occorre dare molta importanza alla possibilità di fruire della pena alternativa in comunità idonee a questo fine (penso alla realtà del mio territorio di Andria). Un ulteriore passo in avanti in tal senso, al fine di evitare, a fronte di condanne brevi, la desocializzazione derivante da una carcerazione di breve durata, privilegiando quindi una finalità retributiva, si è avuto in virtù di quanto previsto dalla legge delega sul processo penale, laddove è stata riformata la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, con la finalità di anticipare l'applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione. L'emergenza carceraria è un problema che da anni sentiamo; innumerevoli fatti di cronaca vedono indistintamente coinvolti detenuti e personale, che a seconda dei casi risultano presunti autori o vittime di fatti illeciti. Ciò è sicuramente manifestazione delle inadeguate condizioni di vivibilità per tutti coloro che ruotano attorno alle strutture penitenziarie. Nessuna violenza può trovare giustificazione né tolleranza; ogni violenza deve essere punita, ma deve anche essere prevenuta. Importante è l'assunzione di personale di Polizia penitenziaria (1.650 agenti e futuri concorsi a bando), così come anche per le figure trattamentali e per i dirigenti penitenziari. Al fine di favorire il trattamento rieducativo del reo, vi è la necessità che gli istituti penitenziari siano dotati di strumenti di controllo automatizzati e sofisticati. Il binomio sicurezza e trattamento è un binomio inscindibile. Anche l'istituto della sorveglianza dinamica, recepito dalle norme europee, che consiste nella permanenza del detenuto fuori dalla cella fino a un massimo di quattordici ore, può essere realizzato solo laddove ci siano sistemi di controllo adeguati, evitando di lasciare un agente a verificare da solo una sezione. Inoltre, mi preme ricordare come molti soggetti privati della libertà presentino patologie psichiatriche, e purtroppo bisogna prendere atto che non sempre ci sono adeguate articolazione ASL per la salute mentale. Bene ha fatto lei, signora Ministra, relativamente al tema della salute mentale in carcere, a mettere in luce la questione relativa alle REMS. Da ultimo, occorre ricordare che, nell'ambito delle pianificazione del *recovery risultano essere diversi gli interventi diretti a migliorare gli ambienti sia per ampliare gli spazi disponibili, sia per realizzare ambienti dedicati al trattamento. A tal fine vi è lo stanziamento complessivo di 132,9 milioni di euro, da destinare alla costruzione al miglioramento di otto padiglioni e alla ristrutturazione degli istituti penitenziari, proprio perché una pena dignitosa deve realizzarsi in strutture adeguate e non certo fatiscenti. Ipotesi come quella del trasferimento dei detenuti stranieri presso il luogo di provenienza è sicuramente una misura che dovrà essere tenuta in considerazione. altresì particolare attenzione alla giustizia riparativa: soltanto mediante la composizione del conflitto tra il reo e la vittima si potrà evitare la recidiva, perché si potrà avviare quel processo di responsabilizzazione del reo e, nel frattempo, mettere il reo a conoscenza delle conseguenze che ha arrecato alla vittima. Solo così il conflitto potrebbe essere riconciliato mediante la presenza di figure specializzate.

qualche notazione su alcuni punti che ritengo siano importanti come tipologia di esperienza. Questa è la mia prima esperienza parlamentare, la mia prima legislatura,

per cui praticamente tutta la parte relativa alle cosiddette pene alternative fu semplicemente - perdonatemi l'espressione - buttata in un cestino.

del Governo. Oggi devo dire che vivo - lo dico convintamente da parlamentare - una situazione completamente diversa.

al clima e alle cose fatte, pur con tutta una serie di criticità e di problematiche che si possono portare dietro (se non si fa niente sicuramente non si hanno critiche, ma quando si fanno le cose automaticamente possono esserci delle critiche, come insegna un vecchio proverbio),

che riguardano la giustizia in questo Paese venivano fatte a costo zero, cioè senza investimenti, senza metterci i soldi, senza avere una prospettiva. Il Ministro ha sempre spiegato che tutto questo dipende

è stato concordato tra il nostro Paese e l'Europa, con a monte delle risoluzioni delle Commissioni parlamentari, votate tra l'altro all'unanimità. quindi di una specie di treno collettivo, che tutti noi abbiamo l'impegno morale e civile, nei confronti del Paese, di mandare avanti nel miglior modo possibile.

la sfida del PNRR, hanno finalmente messo la giustizia al centro, talmente al centro che solo fare l'elenco di tutto quello che è stato fatto, oggi porterebbe via una mezz'oretta, solo per leggerne i capitoli.

e determini conseguentemente un ausilio fondamentale anche per il raggiungimento dei risultati. Non possiamo pensare di avere grandi riforme della giustizia, se non sono accompagnate

la condizione dei nostri penitenziari e tutte le considerazioni che da lei sono state espresse a questo riguardo, rispetto a questo

di vita quotidiana nel pianeta carcere sono direttamente proporzionali alle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria; questo per una banale e semplice constatazione, ossia che vi è un rapporto di causa-effetto tra

il suo comportamento, sempre nell'ambito della normativa e della legge, nei confronti dei detenuti. È banale quanto le sto dicendo,

esprimere questa considerazione. I servitori dello Stato, divisi in Corpi, sono tutti, per quanto mi riguarda, nostri eroi quotidiani; ma se volessimo stilare una graduatoria di quelli che sono sottoposti a condizioni di lavoro più difficili e complicate, io non ho dubbi riguardo al fatto che gli agenti polizia penitenziaria sono veramente quelli maggiormente messi in difficoltà.

agente. Ministro, è sufficiente accedere a qualche penitenziario - e non basta l'esempio del penitenziario di Firenze: le dico che quasi tutti i penitenziari, salvo qualche rarissima eccezione, sono nelle stesse condizioni - per percepire questo grande, grandissimo problema. Ministro, faccio appello alla sua sensibilità. Il corpo degli agenti di Polizia penitenziaria fa riferimento al suo Dicastero, evidentemente, quindi sollecito, per quanto possibile, una maggiore attenzione alle condizioni di vita quotidiana degli agenti, sempre più, peraltro, vittime di episodi di aggressione da parte dei carcerati.

Signor Presidente, colleghi, colleghe, la sua riforma, signor Ministro, qualche cambiamento lo contiene, ma purtroppo l'occasione di operare una svolta storica non è stata Eppure per la crisi così marcata, che mostra clamorose crepe nel sistema della giustizia, si poteva e si doveva fare di più. Due sono le ragioni: un'amministrazione così sfilacciata, che oggi stenta a stare nel cuore delle persone, aveva bisogno di recuperare un umanesimo giudiziario, per evitare tutti i processi degenerativi cui abbiamo assistito; occorreva, inoltre, l'eliminazione totale di quella lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali, che è un limite alla potenziale crescita dell'Italia. La sua riforma, signor Ministro, è stata un compromesso al ribasso, purtroppo. Peraltro è prevalso, come preoccupazione prioritaria, più il problema della efficienza organizzativa della macchina giudiziaria che il tipo di chiusura giudiziale che tende a predominare tra i magistrati penali. L'amministrazione della giustizia in Italia è interessata, in questa fase storica, da importanti riforme, richieste sia dall'interno, per lo stato di degrado e di crisi che il settore vive ormai da decenni, sia dall'esterno, così come è stato anche da lei ricordato, soprattutto dall'Unione europea, nella prospettiva di rafforzamento dell'affidabilità del Paese per la migliore resilienza. Com'è noto, tre sono i capitoli di dette riforme, alcune delle quali già in fase di attuazione. Noi quelle riforme le vorremmo così. La riforma della giustizia civile, per una svolta in favore dei cittadini e degli operatori economici per la garanzia della certezza del diritto; la sicurezza economica nella regolazione delle attività d'impresa e dei contratti; la tutela dei diritti della persona e delle fasce deboli; la realizzazione della Costituzione attraverso una risposta efficace, pronta e sicura alle istanze di giustizia civile, contrattuale, fallimentare e familiare; la riforma della giustizia penale, per un maggiore rispetto dei diritti umani coinvolti nel processo e nell'esecuzione della pena, delle garanzie della difesa in ogni Stato e grado del processo per la lotta ad un esasperato panpenalismo, alla supplenza delle procure, ai difetti o ai ritardi dell'amministrazione attiva, per un riequilibrio del ruolo dell'ufficio di procura nello svolgimento del procedimento penale, con la posizione dei difensori per una moralizzazione dei rapporti tra giustizia ed informazione, magistratura e dell'ordinamento giudiziario per una magistratura più moderna e responsabile, realmente indipendente dalla politica, aperta all'internazionale, per un Consiglio superiore della magistratura effettivamente autonomo dalle correnti, per una valutazione dei magistrati basata sul merito e non sulle raccomandazioni o sulle appartenenze: il il caso Palamara ha insegnato tanto, ma non ha risolto il problema, se ancora nell'ultima settimana il Consiglio di Stato ha decapitato i vertici della suprema Corte di cassazione, annullando le nomine del Presidente e del Presidente aggiunto della Corte di legittimità. Ciò per cui ci batteremo e vorremmo batterci, signor Ministro, è un Paese libero da un condizionamento pesante basato sull'uso della giustizia come strumento di intervento, a volte a gamba tesa, nell'agone della politica.

di fucina della certezza del diritto e dei rapporti giuridici, così come il fatto che i quotidiani, addirittura di fronte ad assoluzioni nel merito, continuino per anni ad adombrare responsabilità inesistenti a carico degli imputati e ripeschino notizie relative a inchieste poi fallite, come se fossero fonti di verità storica assoluta. L'ingegneria reputazionale che segue lo sviluppo delle inchieste finisce per stravolgere il sacrosanto principio della presunzione di innocenza su cui si fonda la civiltà giuridica del nostro Paese. C'è poi un tema importante, ma sempre poco avvertito, Mi complimento con lei perché si è molto soffermata su questo punto, però vorrei dire anche la mia. Restano inalterate le condizioni croniche di sovraffollamento, spazi angusti per un numero davvero eccessivo di persone, come lei ha ricordato: una capienza di 40.000 posti per più di 50.000 persone. Mancano efficaci controlli controlli di sicurezza; sono carenti medici, psicologi, educatori, agenti e mancano percorsi riabilitativi per il rientro nella società. Ci auguriamo che la costruzione di nuove strutture e la diminuzione del numero dei reati per i quali si ricorre al carcere possano invertire una direzione di marcia assurda e poco aderente alla Costituzione. Se al fatto

Un ultimo dato vorrei condividere, signor Ministro. Il 2022 è l'anno del trentennale delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, un momento storico che vide tutta la Repubblica unita per reagire alle offensive della mafia siciliana. Noi avvertiamo ancora oggi e sentiamo nostro quello spirito di trasversalità e di risposta all'indirizzo politico costituzionale che aiutò il Paese a superare brillantemente - oggi possiamo dirlo - una delle più grandi sfide della sua storia. Confidiamo nella sua statura di costituzionalista, tra le più attente studiose dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, per condurre in porto nel migliore dei modi le riforme di cui la giustizia e l'Italia hanno assolutamente bisogno. La lettera che lei ha letto all'inizio del suo intervento è un appello affinché tutto questo si realizzi. Mi auguro che avvenga, signor Ministro, perché essendo stata io stessa vittima di una giustizia lunga, che è durata più di dieci anni senza aver mai riportato condanne in primo grado, posso assicurare a lei e all'intero Senato che sono ferite sanguinanti, che non si chiudono mai per tutta una vita, per cui è importante che lei

moltissimo per questa sua relazione, che giunge al termine di un anno molto complicato, molto difficile per il nostro Paese. Molte sono le tensioni, ma molto è stato anche il il lavoro fatto, rispetto al quale diamo un riconoscimento e un ringraziamento alla sua persona. Ho apprezzato molto la sua determinazione nell'individuare il compito di noi legislatori, che dovrà rafforzare ulteriormente il lavoro sulla giustizia. Non esiste giustizia amministrata in nome del popolo e nel rispetto della legge se non è garantita piena effettività al diritto di accesso alla giurisdizione e al diritto di difesa. di questo legame strettissimo tra giustizia e diritti che parlerò brevemente. L'onestà intellettuale ci porta a riconoscere, purtroppo, che il 2021 non è stato un buon anno per i diritti e per l'uguaglianza in questo Paese. Si è concluso con l'applauso vergognoso di una parte di questa

quelle stesse condotte e quei crimini d'odio che ha ricordato la Ministra nella sua relazione e che hanno alimentato nella storia le peggiori atrocità, unendosi all'indifferenza, alle discriminazioni e alla costruzione dell'altro come un nemico da colpire. Il 2021 è stato anche un anno di moniti, purtroppo rimasti inascoltati dalla Corte costituzionale verso il legislatore. Il Parlamento è fermo, ammettiamolo colleghi. È fermo sul fine vita, è rimasto assolutamente indifferente all'appello della Corte costituzionale nelle sentenze nn. 32 che chiedeva di assicurare tutele e pari dignità ai bambini delle famiglie arcobaleno, bambini diversi, bambini puniti solo per il modo in cui sono nati o solo per i genitori che hanno. Il 2021 è stato, insomma, l'ennesimo anno in cui il Parlamento ha voltato le spalle a tante, troppe domande di riconoscimento di uguaglianza e di giustizia, perché potremmo riorganizzare il servizio giustizia nel modo migliore possibile, ma se le leggi continueranno ad essere insufficienti, se ai giudici si continuerà a chiedere di sostituirsi al legislatore, un legislatore sordo, un legislatore inerte, e il Parlamento continuerà a decidere di non decidere, il legame tra giustizia e diritti sarà sempre più indebolito e sempre più sbilanciato. Il 2021 è stato anche l'anno in cui si è intensificata la barbarie della violenza maschile sulle donne, anche e soprattutto in famiglia. Ho riscontrato nella relazione della Ministra una fortissima attenzione su questo tema, tema, un grandissimo lavoro anche delle tante persone che dentro e fuori dal Parlamento operano per dare dignità a queste donne che chiedono aiuto e soprattutto di essere ascoltate.

Il 2021 è stato anche l'anno in cui abbiamo letto le cronache di momenti molto duri di violenza, come la vicenda del carcere di Santa Maria Capua Vetere, che cito come esempio patologico di quella che, nonostante tutti gli sforzi, resta un'emergenza. Sullo stato delle nostre carceri riconosco a lei, signora Ministra, una fortissima attenzione, anche in accordo e in supporto con la parte più garantista di questo Parlamento, che non ha mai fatto mancare il suo lavoro su questo tema. questo tema. In aggiunta a quello che la Ministra ha ricordato, proprio per dimostrare ciò che ha detto lei, signora Ministra, cioè che il lavoro è stato enorme e quanto lavoro è stato fatto, vorrei citare alcuni passi non citati nella sua relazione. Penso alla questione dei bambini in carcere, con l'adozione del decreto di riparto dei fondi per la realizzazione di case famiglia protette, stanziati nella legge di bilancio del 2021, e anche il rinnovo, per ulteriori quattro anni, della Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti. signora Ministra, a lei va dato atto di aver fatto molto anche su questo. Avanzamenti importanti, che devono però essere sostenuti, monitorati e messi a sistema in un contesto carcerario moderno, con più personale, con percorsi differenziati e con un maggiore investimento sul lavoro e sulla scuola, in carcere e all'esterno. Nella mia attenzione costante al tema delle carceri, sono guidata da un principio molto semplice: chi è detenuto resta anzitutto una persona, una persona che ha più valore delle sue stesse responsabilità. Ce lo insegna l'articolo 27 della Costituzione, che prevede che la rieducazione del condannato non coincida solo con la maturazione della consapevolezza di ciò che si è fatto, ma anche e soprattutto con la preparazione al reinserimento sociale. Su questo vorrei essere molto chiara. Occorre garantire alla persona detenuta una qualità di vita, non solo decente, come dice la relazione Ruotolo, ma che possa permettere al singolo di riappropriarsi della vita di riappropriarsi della vita in tutti i suoi aspetti. Ne ricordo solo uno: la questione dell'affettività in carcere. È incardinato in Commissione giustizia un testo che io chiedo a questo Senato di non dimenticare. Nella sezione

entra in carcere un'intera famiglia. Domandatevi cosa accade ad una madre, ad una moglie, ad un figlio, nel momento in cui l'uomo che ama, la donna che ama, entrano in carcere. Comincia un incubo di orari: l'orario in cui si possono

possibilità di miglioramento della vita di chi ha un detenuto in famiglia, perché queste sono famiglie, non solo private dell'affettività, ma costrette ad un percorso di burocrazia quotidiana durissima, che purtroppo il Covid-19 ha aumentato. Sono certa che troveremo, anche su questo, una modalità di procedere nel segno migliore e sempre nel segno dell'articolo 27 della nostra Costituzione.

per una giustizia vista come una vera e propria infrastruttura democratica, posta al centro dell'attenzione e delle energie di questo Governo, sapendo bene che anche l'erogazione delle somme della Commissione europea per il PNRR è subordinata all'approvazione di riforme di sistema su cui ci siamo davvero spesi. La tenuta del sistema intero, però, è stata messa a dura prova dall'emergenza sanitaria e dalle sue complessive ricadute. I soggetti individuati come responsabili della tenuta dello stesso, in particolare gli avvocati e i magistrati, sono stati attinti da una necessità: quella di adattare lo svolgimento delle attività alle nuove esigenze, a del tutto rinnovate esigenze, con l'impegno non trascurabile di salvaguardare in ogni caso il ruolo e la funzione. Sappiamo che la giurisdizione quale strumento di garanzia e di equilibrio nell'ottica della risoluzione dei conflitti ha rischiato e rischia tuttora di essere sacrificata. La relazione denota una chiara visione di insieme; le riforme denotano una visione davvero ampia, necessaria e funzionale a qualsiasi proposta, soprattutto quella in riferimento all'attuazione dei decreti delegati da adottare in questa fase di *governance* e di attuazione. è tenuto conto del mancato o comunque non adeguato investimento in risorse umane, strutturali, in risorse infrastrutturali, come è evidente anche dalla La crisi della giustizia è un problema che, purtroppo, prescinde dal momento: investe la società, la comunità civile, ai cui margini, ancora una volta, è relegata la tutela della persona, soprattutto se detenuta, come è stato ampiamente documentato, tenuto conto anche delle attuali anche delle attuali condizioni degli istituti penitenziari. Essenziale - nell'esercizio della giurisdizione - è il pieno svolgimento del confronto processuale, ancorato alle garanzie ed espressione di diritti non comprimibili, soprattutto se riferiti ai più deboli, soprattutto se riferiti ai più deboli, ai più fragili. Penso al ruolo di uno degli attori protagonisti, l'avvocatura da cui provengo - anche forte del privilegio di aver avuto in passato la rappresentanza istituzionale per un periodo dell'avvocatura - che nel corso di questi lunghi e difficili mesi ha dovuto resistere, non sempre però riuscendovi, al rischio di una paralisi dell'attività giudiziaria, che ha fortemente inciso sulle irrinunciabili aspettative di tutela L'avvocatura ha dovuto subire le conseguenze di provvedimenti che spesso non hanno ritenuto di dover considerare in adeguata misura la necessità per gli stessi avvocati di accedere in sicurezza agli uffici giudiziari. Un miglioramento

Una considerazione è necessaria, e ha fatto piacere l'evidenza circa l'apporto che la magistratura onoraria fornisce all'esercizio della giurisdizione, anche alla composizione degli stessi consigli giudiziari, al ruolo e alla funzione degli avvocati che ne fanno parte. I problemi che sono venuti fuori dall'analisi sono chiari: la quantità del contenzioso, la qualità delle decisioni, i tempi del giudizio. A titolo esemplificativo, ogni anno sopravvengono in Cassazione più di 30.000 ricorsi civili e 50.000 ricorsi penali, un dato quantitativo unico anche nell'esperienza giuridica internazionale. La qualità delle decisioni è imposta dal ruolo, i tempi del giudizio devono essere tali da rendere la durata complessiva del processo ragionevole, come richiede la Costituzione, e la CEDU ha più volte ricordato che la tempestività e la prevedibilità delle decisioni concorrono a rendere la giustizia conforme ai principi dello stato di diritto e di un sistema democratico. Far quadrare questi elementi - ecco la sfida, che ha un *timing* anche molto stretto - è molto complesso e la situazione attuale è estremamente problematica per le incrostazioni del passato che si sono cumulate. I numeri sono oggi più che mai inarrestabili e questo si riflette anche sugli altri elementi: i tempi del processo civile superano il livello della ragionevolezza, la qualità dei provvedimenti non sempre è all'altezza i contrasti molto spesso inconsapevoli sono diffusi e ricorrenti. Tutto questo dipende da fattori non solo contingenti, ma strutturali, che possono essere letti da una serie di angolature. Come dicevo, la Commissione europea subordina l'erogazione delle somme nel sistema giustizia all'approvazione di queste riforme di sistema e all'attuazione delle stesse, per cui il tema è davvero centrale e i riflessi sono ad ampio raggio nel settore non solo civile, ma in tutte le sue declinazioni; penso all'economia, alla famiglia, al lavoro, ai tanti temi all'ordine del giorno del dibattito - non solo nostro - sulle difficoltà del Paese in tutti i suoi gangli vitali. Le riforme prevedono una serie di deleghe che dovranno essere esercitate; si potenziano gli strumenti in particolare di risoluzione alternativa delle controversie con una nuova cultura anche sociale verso le ADR (*alternative dispute resolution*) da esperire anche con modalità telematiche che devono essere potenziate, che abbiamo visto implementate soprattutto in questa fase pandemica. Fa piacere il passaggio da una fase emergenziale a una fase strutturale delle *best practice* e di tutto ciò che è venuto fuori con successo; un incentivo fiscale, quindi anche premiale, per la mediazione sia civile che commerciale, intervenendo altresì sulla disciplina dell'arbitrato, prevedendo anche l'inserimento di norme in tema di arbitrato societario all'interno del codice di procedura civile. Lo stesso testo reca una serie di modifiche al processo civile di primo grado per migliorare l'efficienza della giustizia, intervenendo sulla disciplina del giudizio di appello, un vero snodo - così come abbiamo più volte documentato - potenziando il filtro di ammissibilità e semplificando la fase di istruttoria del procedimento. la possibilità per il giudice di proporre il cosiddetto rinvio pregiudiziale, ossia di sottoporre direttamente alla Corte la risoluzione di una questione di mero diritto su cui il giudice abbia già sollevato il contraddittorio delle parti, purché sia questione del tutto nuova, di particolare importanza e suscettibile di presentarsi in numerosi giudizi, fonte di gravi difficoltà interpretative: si palesa come una misura estremamente utile. La modifica della disciplina del processo esecutivo, valorizzando le misure di coercizione indiretta e di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile, è un altro elemento fondamentale. con riguardo alle espropriazioni, la possibilità per il debitore di vendere direttamente l'immobile pignorato a un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima: tutti elementi fondamentali che impattano sulla vita delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Le riforme evidenziate introducono altresì misure di riordino e implementazione delle disposizioni necessarie sul processo civile telematico; mi viene da aggiungere anche sui processi ormai telematici e sull'interoperabilità degli stessi: un tema di cui tenere assolutamente conto. Una delle principali missioni del PNRR riguarda proprio la digitalizzazione, con un notevole impegno di spesa: è un'occasione unica. Si interviene quindi sulla disciplina dell'Ufficio per il processo, prevedendo l'istituzione di strutture organizzative analoghe a esso, previste presso la Corte di cassazione e la sua procura generale; introducendo un rito unico applicabile in tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie; prevedendo l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. In conclusione, sono sono note da tempo le relazioni molteplici che legano giustizia ed economia; una giustizia che funziona garantendo attuazione dei contratti e protezione dei diritti; che facilita la vita degli scambi; incoraggia gli investimenti e rende più agevole l'accesso al mercato del credito; favorisce la concorrenza; aumenta - come aumenterà - l'attrattività del nostro Paese nei confronti degli investitori esteri. Sono tutti i temi a cui puntiamo sulla scorta di queste riforme e sull'attuazione delle stesse in via assolutamente prioritaria. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, signora Ministra, approfitto dell'occasione per fare un approfondimento doveroso in merito alla situazione di Foggia e Provincia. Le bombe degli ultimi giorni - ben nove in un lasso di tempo brevissimo -hanno preoccupato, anzi direi scioccato l'opinione pubblica nazionale e internazionale, mentre quella locale lo era già da molti anni. L'aperta sfida allo Stato, le modalità violente e feroci, quasi terroristiche, con le quali agiscono le mafie foggiane destano sgomento, paura profonda e diffuso allarme sociale. Ne hanno parlato i *media* di tutto il mondo, rappresentando una situazione drammatica, nonostante - voglio rimarcarlo - il lavoro costante e penetrante svolto con grande professionalità e sacrificio dalla magistratura circondariale e distrettuale, dalla prefettura e dal personale delle Forze dell'ordine. Ringrazio tutti loro dal più profondo del cuore. Posso affermarlo senza timore di essere smentito: la riforma della geografia giudiziaria del 2012, almeno per ciò che concerne la Provincia di Foggia, ha fallito. Ha fallito completamente con la soppressione del tribunale e della procura di Lucera e quella di altre sei sezioni distaccate, in un territorio che è più grande dell'intera Liguria che ha quattro tribunali, più grande del Molise che ha tre tribunali e simile al Friuli, che ha quattro tribunali. In un territorio del genere, che ha quasi 700.000 abitanti e comprende estese zone impervie funestate dalla presenza di *clan* mafiosi, questa soppressione ha creato un imbuto che impedisce di celebrare con celerità i processi. Ne pendono quasi 13.000 in fase di giudizio. Questo dato, raddoppiato

invece con la concentrazione di tutti gli uffici nella sede foggiana mancano le aule, gli spazi sono insufficienti, gli uffici scoppiano. Insomma, nonostante l'abnegazione dei magistrati e dei dipendenti amministrativi, che ringrazio, la macchina giudiziaria non può funzionare al meglio, anzi direi che è ben lontana da un funzionamento accettabile. Di queste disfunzioni e difficoltà oggettive si avvantaggiano i sodalizi criminali e ne pagano le conseguenze i cittadini, le vittime di reato e tutti gli operatori del diritto. Le soppressioni di tribunali, delle sezioni distaccate e l'accorpamento nell'unica sede di Foggia non solo non hanno portato i benefici ipotizzati dal legislatore del 2012, ma anzi hanno creato un disastro in cui tutti - davvero tutti - ci rimettono, tranne i criminali. Ebbene, se questo è il quadro - e sfido chiunque a dire il contrario - la politica ha il dovere di prenderne atto e di dare risposte concrete. Diversamente le parole di solidarietà giunte da tutti rimarrebbero parole al vento. Io vivo in quel territorio e sento enorme la responsabilità sulle mie spalle, ma dovremmo sentirla tutti noi e dovremmo avvertire tutti la necessità di prendere immediatamente provvedimenti drastici. Il procuratore nazionale antimafia, dottor Cafiero de Raho, ha parlato più volte della situazione foggiana come di una vera e propria emergenza nazionale. Ebbene, visto che siamo in una situazione di emergenza che preoccupa tutto il mondo, occorre avere il coraggio e la forza di prendere decisioni eccezionali, senza farsi condizionare dal *totem*, dal *moloc* dell'intangibilità della geografia giudiziaria o - per esempio - dell'attuale disposizione e ubicazione dei commissariati di Polizia di Stato. Nello specifico, come MoVimento 5 Stelle, abbiamo chiesto alla ministra dell'interno di rafforzare considerevolmente il numero delle Forze dell'ordine in provincia e di elevare i commissariati di San Severo e Cerignola a strutture di primo livello. Sul versante giudiziario chiediamo da tempo che vengano istituiti almeno un altro tribunale e almeno una sezione distaccata che possano coprire le zone Sud e Nord di questa estesa Provincia. Inoltre il MoVimento 5 Stelle, a mia prima firma, ha depositato, fin dall'agosto del 2018, un disegno di legge per l'istituzione a Foggia di sezioni distaccate della corte di appello di Bari, (DDA) e del tribunale per i minorenni. Analogo disegno di legge è stato presentato alla Camera nel 2021 dalla collega Giuliano. Le ragioni sono ovvie e sono diffusamente illustrate nella relazione del mio disegno di legge, a cui rimando e non ripeto qui soltanto per ragioni di tempo. Infine, nelle more dell'auspicata

che si occupano stabilmente ed esclusivamente di reati di stampo mafioso in quella Provincia. Ciò renderebbe ancor più proficuo il loro lavoro e quello della Polizia giudiziaria perché presidierebbero meglio il territorio, evitando perdite di tempo a fare la spola tra Bari e Foggia. Se a queste nostre proposte, fattibili e di buon senso, non seguiranno atti concreti da parte di chi ha responsabilità legislative, organizzative e di governo, vorrà dire che le belle e accorate parole pronunciate in questi giorni da tutti sono state un mero vuoto e insopportabile esercizio di stile. In tal caso i cittadini della mia meravigliosa e sfortunata provincia ci giudicheranno. *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signora Ministra, signori Sottosegretari, stimati e cari colleghe e colleghi, ho ascoltato con molta attenzione la relazione della signora Ministra devo dire che in gran parte è condivisibile. Ovviamente ci sono dei distinguo che io cercherò di fare. Anzi, avviso che, avendo poco tempo a disposizione, occuperò

in maniera corretta ed esaustiva i grandi temi che affliggono purtroppo questo settore. È evidente che il settore della giustizia - lei, Ministra, lo ha esposto molto bene - ha bisogno di una revisione profonda, per tutto quello che sta accadendo ed è accaduto negli ultimi anni. Sappiamo quali conseguenze dannosissime sono derivate al nostro Paese da una gestione non ottimale del settore, soprattutto negli ultimi anni. La lettera che lei ha letto, sicuramente toccante nella sua tragicità, non rappresenta che uno degli aspetti deteriori del nostro sistema. Si pensi a quella persona che purtroppo ha deciso di togliersi la vita dopo aver affrontato un processo durato dieci anni, conclusosi con un'assoluzione in primo grado e una condanna in secondo grado;

autorizzando qui un arresto. E poi, dopo cinque anni di processo e due anni e mezzo di carcere, è stato assolto perché il fatto non sussisteva. Ecco, sono questi i temi che dovremmo prendere in considerazione. A proposito di quello quello di cui parlavo in precedenza, non possiamo non sottolineare la necessità di mettere mano e di rimediare anche al fatto dell'appellabilità della sentenza assolutoria di primo grado, perché, se è vero che la condanna deve arrivare quando c'è la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, non si capisce per quale motivo, se un magistrato con le sue competenze è arrivato alla conclusione che una persona è innocente, ci debba essere la possibilità di riprendere in mano tutta la vicenda. Si deve andare forse alla ricerca di chi invece legga la vicenda in maniera diversa? maniera diversa? Chi frequenta le aule giudiziarie sa perfettamente che qualsiasi vicenda presenta due facce differenti. a una ci si deve attenere. E noi crediamo nella preparazione della nostra magistratura. Io ripeto sempre che, facendo l'avvocato, devo continuare ad avere fiducia estrema nella magistratura, perché altrimenti non potrei fare l'avvocato; preferirei andare in tabaccheria a comprare una schedina del SuperEnalotto. Invece mi affido alla magistratura, conoscendo la preparazione e il livello altissimo che noi abbiamo; ma il sistema va cambiato. In questo senso debbo dire che ovviamente stiamo facendo i conti da anni con i cronici ritardi nella definizione dei tempi del processo. I cittadini da noi si aspettano molto in questo senso, ed è evidente che si aspettano molto. Da anni purtroppo ancora non siamo riusciti a dare loro una risposta concreta ed esaustiva.

durante il cammino si aggiusta il carico. È un vecchio proverbio sardo e la saggezza popolare talvolta aiuta anche nella quotidianità della vita. Probabilmente sarà necessario mettere mano ad alcune cose. Ho parlato poco fa dell'appellabilità delle sentenze assolutorie di primo grado, per citarne soltanto una. Mi permetta, signor Ministro, perché, a causa dell'età che ormai avanza, non vorrei dimenticarmene. Lei ha citato il caso Regeni. Mi permetto di aprire una parentesi rapidissima: credo sia necessario che il Ministero si occupi in maniera un po' più fattiva anche della vicenda di Chico Forti, che ormai è un fatto notorio che deve essere affrontato in maniera determinata, perché dobbiamo riportare a casa una persona che evidentemente è stata vittima di un errore giudiziario. Si giudiziario. Si è parlato della carenza di personale, si è parlato della carenza di spazi adeguati e di risorse umane e strumentali: in tutti e tre i settori c'è davvero tanto da fare.

Debbo dire che è stato sì avviato un percorso, ma voglio sottolineare che quel percorso era stato avviato dal ministro Orlando, che aveva finalmente riaperto i concorsi in magistratura magistratura e aveva anche dato avvio alle procedure concorsuali per il personale amministrativo. Voglio anche sottolineare un'altra cosa: ciò non basta perché, finché non c'è certezza dell'organico al completo, non avremo la possibilità di avere una giustizia in tempi certi e determinati. È una vicenda della quale dobbiamo occuparci immediatamente. Credo che si stia già facendo molto e bene ha fatto la signora Ministra a sottolineare che di recente è stato bandito un concorso per 500 posti. Debbo anche dire che i risultati non sono certamente incoraggianti, almeno per quel che si sente dire; pare che non siano molto incoraggianti, ma a mio parere dobbiamo insistere in quel percorso.

i femminicidi, che purtroppo nel 2021 sono stati 109; non sono numeri, ma sono donne uccise, spesso mamme.

di intuire e prevenire le conseguenze anche fatali, e ha invocato una profonda riforma delle procedure e dell'organizzazione giudiziaria. giudiziaria. Ministro, lei ha fatto anche un cenno - e questo è l'oggetto principale del mio intervento - a un disegno di legge approvato in Consiglio dei ministri

disegno di legge è volto a rafforzare gli strumenti di prevenzione anche a completamento di quanto già previsto dal codice rosso, che anche noi abbiamo votato ma che nell'applicazione ha dimostrato di richiedere qualche aggiustamento. Del resto c'è anche un *vulnus*, un buco, nella riforma del processo penale come denunciato nel mese di dicembre dalla procura di Tivoli - rispetto a quanto accade nel momento in cui si arresta colui che viola il divieto di avvicinamento ai luoghi di frequentazione della vittima. Magari il giorno dopo l'arresto viene processato per direttissima, ma viene rimesso in libertà nella condizione vieppiù di nuocere alla vittima. vostro disegno di legge, con undici articoli se non erro, andava a colmare anche quest'aspetto che non è né marginale né banale.

e che va anche a migliorare aspetti della riforma del processo penale, perché contiene misure stringenti per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, è stato

per chi viola il suddetto divieto di avvicinamento alla vittima, in modo da prevenire più efficacemente il rischio di condotte violente reiterate; inoltre, al di fuori dell'arresto in flagranza di reato si potranno applicare le misure cautelari. Signor Ministro, intanto dov'è finito questo disegno di legge? Il nodo è - lei lo ha detto e lo sa, ma purtroppo lo sappiamo tutti, per i casi di cronaca - che bisogna rafforzare l'arresto obbligatorio in flagranza, per evitare quello che dicevamo, cioè il processo per direttissima e le

in Parlamento? Perché di fronte all'evidenza di questo fenomeno emergenziale e drammatico non si è proceduto? Perché il Governo non ha voluto emanare un decreto-legge, invece che un disegno di legge, che notoriamente

*(Applausi)*. Non c'è tempo da perdere: non si perda tempo! Lei ha ricordato Paolo Borsellino e mi permetto di ricordare, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, che oggi di Paolo Borsellino ricorre la data della nascita. È quindi una sorta di compleanno: onore a lui e alla sua memoria. Signor Ministro, la prego: ormai avete scelto la strada lunga del

riforme necessarie per il Paese: prima di tutto per il Paese e per i cittadini. Certamente molto resta da fare, ma le scelte fatte sul processo civile e sul processo penale sono positive e importanti e non si limitano - come lei giustamente ha ricordato nella relazione - a intervenire sulla velocità dei processi, agendo anche sulla qualità dei processi e del diritto. Ci sono, nella relazione e nel lavoro svolto quest'anno, alcune questioni che ci sta a cuore sottolineare, condividendone ovviamente l'impostazione. La prima è certamente la scelta di intervenire molto sull'organizzazione della giustizia. L'investimento, consentito anche dal PNRR, sull'organizzazione, sulla digitalizzazione, sulle infrastrutture della giustizia è decisivo e fondamentale. Le assunzioni per l'Ufficio del processo, insieme alla promozione e all'incentivazione dell'utilizzo di strumenti alternativi alle controversie, in particolare la mediazione civile, sono scelte decisive per migliorare. La seconda questione riguarda il penale. Voglio sottolineare una cosa che per noi ha una grande importanza: con queste riforme si comincia a invertire una tendenza, si esce dalla logica del buttare via le chiavi, si prova a tornare alla Costituzione. Al di là e oltre la giusta depenalizzazione dei reati bagatellari, è importante che, nella pratica, si stabilisca il principio che il carcere non è l'unica scelta per sanzionare i reati. Nella norma della riforma del processo penale e, ancora di più, nella relazione si insiste sulle pene alternative, sulla messa alla prova, sulle pene risarcitorie. È giusto. Questi sono gli strumenti per recuperare la funzione riabilitativa della pena. Sappiamo bene che, per andare su questa strada, servono ulteriori investimenti, assunzioni nelle aree trattamentali, riconoscimento delle professionalità. Servono concretamente norme

continuo a pensare che questa sia la via maestra per superare l'emergenza, che anche lei, Ministro, sottolineava, della sovrappopolazione carceraria. È chiaro, però, che devono essere assunte

il 31 marzo e oltre la fine dell'emergenza delle misure che abbiamo messo in campo per ridurre i disagi all'interno del carcere a causa del Covid-19. Come terza questione, accanto a ciò, signor Ministro, lei ha avviato una riflessione, per noi di straordinaria importanza, sulla giustizia riparativa. una riflessione che mette al centro le vittime, spesso dimenticate, e che mette il reo di fronte alle proprie responsabilità. Anche su questo spero si possa rapidamente andare oltre la teoria o le sperimentazioni episodiche, per mettere concretamente a terra l'attivazione di tale strumento. Non è una critica, anzi: c'è il riconoscimento di una riflessione importante che, al più presto, deve produrre soluzioni. Infine, le recenti sentenze della Corte costituzionale e delle Corti europee portano il Parlamento

penitenziario e dell'ergastolo ostativo per noi deve muoversi in questo spazio stretto: garantire il rigore per impedire a chi non ha spezzato i fili con le mafie con le mafie di poter avere alcun beneficio, ma, dall'altra parte, mettere lo Stato nelle condizioni di riconoscere il cambiamento. Ministro, l'esperienza di quest'anno dimostra che, se si sta al merito e si esce dalle contrapposizioni ideologiche, anche sulla giustizia, le riforme si possono fare, non contro qualcuno, ma nell'interesse dei cittadini e del Paese.

di questo la ringrazio. Penso che le proposte dettagliate della relazione vadano sostenute e aiutate, e questo lo mettiamo da parte. Quello che invece voglio sottolineare, per il futuro e non per guardare indietro, è la necessità delle riforme che mancano e che - secondo noi - da trent'anni sono essenziali.

è anche una questione di efficacia. Lei ha ricordato il tema della fiducia. Noi viviamo in un momento in cui i cittadini non hanno fiducia nella giustizia, ben che vada ne hanno paura e pensano - giustamente e peraltro in molti casi - che, se per caso finiscono in una delle maglie della giustizia, si ritrovano in un tunnel kafkiano dal quale non escono più, con tutta una serie di danni reputazionali, familiari ed emotivi che nessuno ripagherà mai, e ripeto: nessuno ripagherà mai. delle carceri lei ha parlato di sovraffollamento, ha dato le cifre, che - ahimè - condivido con la mia amica Rita Bernardini.

attualmente positivi, per cui siamo in una situazione che richiederà non solo l'attuazione degli impegni che lei ha preso e le riforme avviate, ma forse anche un qualche intervento di emergenza.

Mi riferisco ovviamente ai temi che riguardano la separazione delle carriere - ad esempio - la responsabilità civile dei magistrati, l'obbligatorietà dell'azione penale; insomma i problemi di fondo creati ben prima che lei arrivasse, ma che penso le toccherà con molta difficoltà cercare di sbrogliare. Ogni giorno i cittadini ne sentono una: ieri era il grande scontro -

e penso che sia questo uno dei motivi della sfiducia dei cittadini, che sento palpabile, perché tra questo e

Questi temi, che la maggioranza non può affrontare, saranno oggetto dei *referendum* chiesti dai Consigli regionali e da una parte delle firme del partito transnazionale.

Sono temi divisivi da trent'anni e, se li vogliamo superare in un modo o in un altro, non si aspetti di trovare una larga maggioranza, perché non sarà affatto così. penso che nella costruzione di tutta questa vicenda anche la la possibilità di depenalizzazione dei reati minori sia una strada importante; in particolare penso alla legalizzazione della *cannabis*. Un terzo dei detenuti è recluso non per droga, eroina, mafia o non so cosa, ma

questo Parlamento è sempre intento ad aggravare le pene, ad inventare nuovi reati, nuovi reati, come se non bastassero. Non è esattamente così come la vedo e come la vediamo noi. Avrà davanti a sé un anno piuttosto difficile anche riguardo all'Europa e alle riforme che si aspettano.

né in politica né nella vita personale: se creiamo un vuoto, qualcuno lo riempie e già sappiamo come potrebbe andare a finire. *(Applausi)*.

Siamo usciti dal terrapiattismo di qualche tempo fa, di qualche Governo precedente, di qualche Ministro che l'ha preceduta e finalmente siamo entrati in una nuova epoca. Questo dobbiamo dircelo. Siamo entrati in un'epoca copernicana: abbiamo scoperto che è la terra che gira intorno al sole e siamo ritornati a parlare nel modo dovuto di diritto e di problemi che affliggono questo Paese e rivestono al suo interno un'importanza fondamentale. L'Europa ci ha imposto delle riforme, a fronte dei prestiti che, diversamente, non arriverebbero. Lei, giustamente, può annoverare, quali risultati ottenuti e concreti, la legge delega sulla riforma del processo civile e penale e il decreto legislativo sulla crisi di impresa, che introduce delle novità dal punto di vista della negoziazione ed evita forse procedure fallimentari inutili. Ha raggiunto questi obiettivi attraverso commissioni di studio, con un ampio confronto in Parlamento, con un'ampia maggioranza, con una complicata maggioranza. Viviamo in un'epoca di complessità: le banalizzazioni sono facili, mentre le complessità sono difficili, e dobbiamo ricercare la complessità per migliorare noi stessi. Mi rendo conto che il lavoro è stato tanto. Giustamente, come diceva la collega Modena stamattina, si è prodotto molto in questo periodo, in questo anno e mezzo. Ho una memoria abbastanza breve e labile, che mi tradisce facilmente,

visione tipica di chi è giudice costituzionale rispetto a quella che possa essere la funzione dell'ufficio del processo. Io ritengo, però, che questo istituto sia un po' difficile da pensare nei tribunali. Immagino che i giudici onorari saranno coloro i quali scrivono le sentenze per i giudici togati: non vorrei che fosse così, ma, nei fatti, in parte è così. Siamo in un Paese in cui esiste un arretrato o una pendenza di circa 4 milioni di processi (oltre 3 milioni di processi civili e oltre un milione di processi penali in abbiamo un arretrato spaventoso e 270.000 avvocati, il cui reddito è inferiore ai 50.000 euro per l'80 per cento (questi sono dati del Censis, quindi sono un esempio di *welfare* sociale del quale bisogna cominciare a ragionare), di circa 9.000 giudici ordinari, come lei questa mattina ci ha ricordato. Eppure, i problemi della giustizia, anche rispetto a quanto diceva chi mi ha preceduto, in un intervento di livello assolutamente politico, assolutamente politico, sono sempre gli stessi sono enormi, giganteschi, in questo Paese. Rispetto a questi, è vero che possiamo anche pensare di ridurre del

del codice di procedura civile o non facendo l'udienza di precisazione delle conclusioni abbiamo risolto il problema della durata del processo civile. Non è che nel processo penale risolviamo il problema, se non affrontiamo i problemi dell'imbuto del secondo grado di giudizio.

nei Paesi anglosassoni e secondo sistemi più civili e collaudati, non sono appellabili, salvo il sopraggiungere di fatti nuovi,

revisione di legittimità, affidata alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 606 del codice di procedura penale, che possiamo tenere come esempio di temperamento del principio di non appellabilità delle sentenze di proscioglimento.

Questo è il principio alla base di tutti i trattati internazionali, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Signor Ministro, altre persone la stanno distraendo in questo momento - immagino per ragioni ben più importanti delle mie - però è questo il tema,

di impugnazione per il pubblico ministero, perché non discende nemmeno dall'articolo 112 della Costituzione, e l'ha chiarito la Corte costituzionale nel 2020, in una sentenza di cui anche lei

anni fa, proprio oggi, moriva ad Hammamet Bettino Craxi, io dico da esule. Visto che oggi stiamo parlando di giustizia, ricordo che non abbiamo ancora risolto quella pagina importante della giustizia *(Applausi)* che è stata la vicenda di Tangentopoli che è stata anche la vicenda recente di colui che si è suicidato alla fine dello scorso anno, Burzi. Al contrario, preferiamo

penale: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Ma quando mai? Sono nove parole che hanno distrutto la giustizia.

non posso che rinnovare la mia personale convinzione che il suo sia stato un lavoro importante e la invito a proseguire con la stessa serietà e concretezza nel lavoro che sta svolgendo.

una lettera che ha voluto leggere a quest'Assemblea; è stato importante, lo abbiamo apprezzato, per non dimenticare mai che la giustizia è una corda profondissima nel cuore di ogni essere umano, e noi a quel desiderio di giustizia siamo chiamati, ciascuno nel suo ruolo e nel suo compito, a dare soddisfazione. Lei ha dato atto della necessità di intervenire con urgenza di fronte agli ultimi inquietanti fatti di cronaca giudiziaria, che hanno minato la fiducia verso la magistratura. Ha parlato nella sua relazione della necessità di ricucire la fiducia dei cittadini verso la magistratura;

Non voglio dimenticare quanto lei ha affermato in relazione alla necessità di intervenire sulle strutture carcerarie, sul supporto agli uomini e alle donne della Polizia penitenziaria. Mi permetto di accennare, Ministro, anche alla necessità di rivedere - e di farlo il prima possibile - alcuni aspetti della normativa di emergenza, che limitano - in alcuni casi anche pesantemente - il diritto alla difesa e al contraddittorio. Credo che ormai si possa decidere di superare quei limiti. Ci sono degli aspetti, che lei ha particolarmente enucleato, in materia di riforma del processo di famiglia. Abbiamo lavorato insieme sulla riforma del processo di famiglia e credo che il lavoro che ne è uscito sia buono, interessante e con delle belle prospettive. Lei ha giustamente iniziato l'argomento parlando di femminicidio, ma mi permetta di dirle, Ministro, che il femminicidio non è

un papà di Napoli, che mi scrive: «Buongiorno senatore, sto affrontando una battaglia da dieci anni contro false accuse di *stalking* e maltrattamenti. Ho subito due processi, in entrambi sono stato assolto. Il tribunale aveva disposto affido condiviso, ma la Corte d'appello ha imposto affido esclusivo, nonostante abbia superato due consulenze tecniche per la valutazione della mia capacità genitoriale. Se può aiutarmi, le sarei grato. Un papà distrutto. 23 giugno 2021». Stefano, un papà di Nuoro, che mi scrive: «Perdonatemi se mi rivolgo a voi, ma è da quasi un anno che non vedo mio figlio. È possibile che una madre con un figlio di quattro anni spariscano dalla faccia della Terra? Il piccolo è stato portato in Bielorussia dalla madre e, nonostante il tribunale locale abbia ordinato il rientro, ai sensi della Convenzione dell'Aia, la madre si oppone e nessuno fa nulla. Vi prego, aiutatemi». Francesco, un papà di Prato, «Buongiorno senatore, vorrei parlare con lei. Sono un papà separato, ho ricevuto una sentenza punitiva. Vorrei solo vedere più spesso mio figlio, ma ora lo posso vedere solo un giorno a settimana. Vorrei pagare il giusto per mantenerlo e non un mantenimento folle. Dovrò dormire in macchina, perché non potrò più avere una casa in affitto. La prego, mi chiami». Anna, una nonna di Milano: «Buongiorno senatore, sono una nonna che non vede il proprio nipote - abita a 500 metri da casa mia - ormai da mesi e anche mio figlio non riesce più a stare col suo bambino di tre anni, nonostante l'ordine del tribunale. Dopo mesi e mesi di processi inutili, i soldi sono finiti e mio figlio è disperato e sfiduciato, non sa più cosa fare e io sono molto preoccupata. La prego, senatore, ci aiuti.» Queste sono storie di vita vissuta, vissuta, sono fatti; noi, di fronte a questi fatti, abbiamo cercato, con la riforma del processo civile, di dare qualche risposta, ma finché non interverremo con un affido davvero condiviso e con una formazione di magistrati, avvocati e altri operatori che sia davvero davvero rispettosa dell'affido condiviso non usciremo da questo *cul-de-sac*. Segnalo Ministro, che è opportuno evitare nel processo di famiglia logiche di contrapposizione tra mamma e papà, tra marito e moglie; non va alimentata la conflittualità endofamiliare, ma promossa una logica di alleanza, non di demonizzazione dell'altro, altrimenti a farne le spese saranno sempre i bambini. Lei ha detto parole che mi sento di condividere e sottoscrivere, oltre che con la penna, anche con il cuore. Ha detto che la giustizia non si nutre di odio, ma ricerca la verità e la cura dei rapporti. La giustizia deve saper unire, più che dividere: questo vale a maggior ragione nel processo di famiglia, che ancora oggi è contenzioso e non può essere figlio delle ideologie. La prego, Ministro, ripeto: il femminicidio è diritto penale, è un'altra cosa; il processo civile e il processo di famiglia non devono essere frutto della demonizzazione reciproca. Ci sono altri argomenti, Ministro, che ci preoccupano, perché impattano sempre sui più deboli, sui più fragili e sui nostri bambini. Quanto accade in in un abuso del processo di famiglia accade anche in altri ambiti. Abbiamo già parlato, con la lettera che ho letto prima, della sottrazione internazionale dei minori, una piaga che purtroppo in Italia non accenna ad arrestarsi. È necessario intervenire e sostenere questi genitori, che non sempre sono maschi pericolosi e paternalisti o - peggio ancora - patriarcali, ma molto spesso sono mamme, che hanno subito la sottrazione del loro bambino, spesso portato dai papà nei Paesi islamici. Bisogna intervenire e sostenere, eventualmente anche con un gratuito patrocinio, le immense spese legali che devono essere sostenute all'estero. Di fronte a tutto questo quadro internazionale, abbiamo con preoccupazione notato l'avanzare di una giurisprudenza creativa, che, nonostante i chiari e precisi arresti della corte suprema di cassazione a sezioni unite e della Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2021, per la legittimazione indiretta di una pratica barbara, inaccettabile, indegna di un Paese civile e contraria a qualsiasi forma di dignità della donna. Mi riferisco all'utero in affitto. Non possiamo legittimare, né *ex ante* né, peggio ancora, *ex post*, una pratica che espone la donna a essere considerata meno di un'incubatrice vivente. Non possiamo permettere che i bambini siano comprati su Internet, che siano scelti da catalogo in base alle caratteristiche fisiche dalla loro genitrice e poi

una moratoria internazionale dell'utero in affitto. Serve che l'utero in affitto sia riconosciuto dal nostro Paese come reato universale. Oggi non è così. Oggi la condotta di chi ricorre alla pratica dell'utero in affitto all'estero non è punita, perché non rientra tra i reati punibili, se commessi all'estero. Ci sono molti altri temi che vorrei affrontare. È in corso di esame alla Camera un disegno di legge già approvato al Senato che mira a prevenire l'autolesionismo e a trasformare l'istigazione all'autolesionismo in reato. Oggi non è così: i nostri bambini e i nostri ragazzi,

all'istigazione all'autolesionismo, insomma, a pericoli assoluti per la loro incolumità. Anche su questo dobbiamo intervenire, non possiamo tacere.

Che di conseguenza la collaborazione è più importante della competizione». Con queste parole del filosofo e matematico inglese Russell apro il mio intervento oggi in Aula per sottolineare e invitare tutti i presenti a riflettere su quanto sia importante la condivisione di intenti per raggiungere risultati importanti. Il Governo di cui facciamo parte è nato in una situazione eccezionale e ha unito sotto lo stesso tetto una pluralità di soggetti con convinzioni e con idee molto distanti tra loro, talvolta antitetiche. Lo ha fatto in nome della gestione dell'emergenza in cui tutti siamo coinvolti e per garantire anche la realizzazione delle riforme indispensabili al bene del Paese. I risultati raggiunti sarebbero stati impossibili, se non vi fosse stata la volontà congiunta di superare i contrasti per arrivare a soluzioni condivise. Governo di emergenza non vuol dire, però, che le scelte e le decisioni prese siano state affrettate e superficiali. Al contrario, è stato importante lavorare con impegno e con attenzione nella ricerca di soluzioni mediane che mettessero tutti d'accordo in nome del più alto interesse pubblico. Di questo *modus operandi* sono stata testimone nei lunghi lavori parlamentari, per arrivare arrivare all'approvazione della riforma della giustizia, che personalmente ho seguito come Capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Commissione giustizia. Per questo ringrazio la ministra Cartabia, che ha saputo conciliare le varie istanze delle forze politiche. Ci tengo a ringraziare anche i miei colleghi, che hanno dimostrato di saper mettere da parte le differenze per valorizzare gli obiettivi comuni. Le riforme del processo civile e del processo penale hanno permesso di imboccare strade virtuose per accelerare i tempi della giustizia e dare così competitività all'Italia e garanzie ai cittadini. Si è scelto di investire nelle risorse umane, proseguendo sulla strada tracciata dal Governo Conte II, rafforzando l'organico e investendo risorse ingenti nell'innovazione più rilevante, costituita Migliaia di giovani giuristi sono stati selezionati per essere destinati agli uffici giudiziari in ausilio al lavoro dei giudici; molti altri invece continueranno a essere scelti tramite i prossimi concorsi pubblici. Ci sono state assunzioni di nuovi giudici e di nuovi funzionari. Inoltre quest'anno finalmente possiamo dire di aver avviato la stabilizzazione di migliaia di magistrati onorari, che per anni hanno prestato il loro indispensabile servizio senza le tutele lavorative più basilari, come la malattia, la maternità o le ferie. Con la riforma del processo civile si è puntato a valorizzare e a perfezionare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (i cosiddetti ADR, Alternative dispute resolution) al fine di ridurre il carico dei tribunali e di incentivare soluzioni consensuali di risoluzione dei conflitti. Importanti incentivi fiscali per tali procedure sono stati pensati come stimolo al maggiore utilizzo e per i non abbienti è stato il garantito il patrocinio a spese dello Stato anche per le procedure extragiudiziarie. L'introduzione del nuovo tribunale della famiglia si è posto come una risposta urgente al problema pressante dovuto ai troppi casi di violenza sui minori e sulle donne. Nell'ambito del processo penale, la legge di riforma ha puntato su interventi volti a diminuire i casi di ricorso al carcere come unica soluzione punitiva, puntando su misure alternative alla pena come la sospensione del procedimento con la messa alla prova dell'imputato, che ha dato ottimi frutti nel sistema penale minorile già dal 2015. La giustizia riparativa è stata introdotta in ogni stato e grado del procedimento, nella convinzione che possa garantire un rimedio dell'offesa e una maggiore attenzione alle vittime. Per quanto riguarda poi la prescrizione, che da sempre è un tema al quale il MoVimento 5 Stelle ha dedicato molta attenzione, è stata confermata la riforma del 2019, che ne blocca il decorso dopo la sentenza di primo grado. Il correttivo dell'improcedibilità, pensato dal Governo e inizialmente irricevibile da parte del MoVimento 5 Stelle, è stato in conclusione accolto, proprio perché si è scelta ancora una volta la strada della mediazione e il risultato è stato il frutto di un punto d'incontro. Un passaggio obbligato è quello sulla situazione delle strutture penitenziarie, che è stata esasperata dalla pandemia. Condivido appieno quanto sottolineato dalla ministra Cartabia nella sua relazione e ritengo sia indispensabile agire con investimenti ingenti per ridare dignità ai detenuti e risolvere problemi annosi come il sovraffollamento, ma anche per mettere finalmente in campo misure di sostegno psicologico e di formazione specialistica per tutto il personale e soprattutto per la Polizia penitenziaria. Il tema della salute mentale in carcere è fondamentale per garantire che la pena rispetti i dettami Quello che noto con rammarico, però, è che nella sua relazione, ministra Cartabia, non abbia in alcun modo citato la necessità di intervenire con una riforma della geografia giudiziaria. Per questo, concludendo, vorrei porre l'attenzione sul tema. La riforma della geografia giudiziaria del 2012, com'è noto, ha operato una radicale riduzione degli uffici giudiziari. Le critiche degli operatori del settore hanno da tempo superato i commenti positivi e, a distanza di quasi dieci anni, i prospettati vantaggi in termini di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli uffici non hanno dato i frutti sperati. A farne le spese, in nome del risparmio, è stato il rispetto del principio di prossimità e del principio di eguaglianza nell'accesso alla tutela dei diritti. Nel concreto, in molti territori, a fronte della riduzione della spesa pubblica, si sono registrati un impoverimento in termini di servizi per la comunità e un aggravio di oneri per l'utenza. Si pensi a tutte quelle realtà che scontano difficoltà di collegamento dovute ad esempio alla carenza di trasporti pubblici o infrastrutture; si pensi alle aree interne, Ministra, che pagano la lontananza dai grandi centri urbani e in termini di distanza dai servizi. A questo si aggiunga la situazione di molti territori. Vorrei ricordare in quest'Aula un caso unico in Italia, che a mio parere richiede un intervento ancora più urgente, quello del soppresso tribunale di Sala Consilina, lo storico tribunale del Vallo di Diano, in Provincia di Salerno, che due primati negativi: è l'unico tribunale ad essere stato accorpato ad un tribunale più piccolo sia in termini di carico di lavoro, sia in termini di dipendenti; ed è l'unico tribunale ad essere stato accorpato a quello di un'altra Regione (di Lagonegro, in Basilicata). La conseguenza è che i cittadini e gli operatori del settore sono costretti a recarsi da una Regione all'altra, ossia dalla Campania alla Basilicata. In secondo luogo, vorrei ricordare che la competente corte d'appello è quella di Potenza, anziché di Salerno. Concludo, signora Ministra, augurandomi vivamente che il tema descritto non passi in secondo piano e si trovino il modo modo e il tempo di affrontarlo al più presto. Lo chiedono a gran voce i cittadini e gli operatori del settore, al cui appello mi Dichiaro chiusa la discussione. Comunico che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, dal senatore Balboni e da altri senatori, n. 2, dai senatori Lannutti, Giannuzzi, Lezzi, Moronese,

Presidente, ringrazio tutti i senatori e le senatrici innanzitutto per la pazienza nell'ascolto della lunga presentazione della relazione introduttiva, per il ricchissimo dibattito che ne è seguito e anche per le parole di apprezzamento, non tanto per me, quanto per il lavoro svolto, che a mio parere davvero avvicina a importanti risultati, che tornano a portare la giustizia al centro delle riflessioni del dibattito pubblico, come dev'essere. In queste repliche (anche per non farmi rimproverare più dalla senatrice Bonino, che mi ha detto di essere stata troppo puntigliosa), ho pensato di raggruppare

gli altri), in direzioni diverse e sottolineando aspetti diversi, si sono concentrati sul carcere e non è un fatto casuale, perché è davvero una delle emergenze che si stanno imponendo in modo sempre più evidente nel nostro Paese.

all'osservazione in cui si è sottolineata una mia disattenzione nei confronti di alcuni aspetti della vita del carcere a favore di altri. altri. Rispondo, innanzitutto, con alcune parole che ho usato nella relazione e che forse sono la testimonianza più evidente di ciò che per me è una convinzione profonda e che cioè, riguardo al carcere, non ci può essere un atteggiamento che contrapponga le esigenze dei detenuti a quelle della polizia penitenziaria e dell'altro personale che ci lavora. Lo abbiamo detto e lo avete ripetuto in tanti: ogni ogni miglioramento di vita all'interno delle case di reclusione e del carcere in generale rende più dignitosa la vita di tutti, stempera le tensioni, abbassa i motivi di attrito che possono esserci. Tutti chiedono in modo convergente - non è un caso - di

Credo non ci sia la possibilità di scindere i due profili e che dobbiamo imparare a superare la logica della contrapposizione degli opposti.

La polizia penitenziaria svolge un compito complesso e delicatissimo, ai miei occhi ancora troppo poco conosciuto. Oltre all'esercizio della tradizionale funzione di vigilanza e di custodia, la polizia penitenziaria è quotidianamente accanto al detenuto e deve essere sostenuta da un'adeguata e costante formazione. In questi mesi ho raccolto molte testimonianze che raccontano quanto sia stata decisiva la presenza di un agente per segnare una svolta nella vita di un detenuto. La scorsa settimana ero in un carcere minorile a Milano, dove si presentava un libro - per chi è interessato, si intitola «Ero un bullo» un giovane di periferia, con un passato criminale tra carcere minorile e rieducazione in comunità. È una storia di quelle in cui si conferma che i nostri Costituenti non avevano solo delle visioni; una di quelle storie di successo che lo ha portato poi a laurearsi e a diventare lui stesso educatore per i suoi compagni. Ebbene, in quella storia uno dei ruoli decisivi, non l'unico, è stato quello del brigadiere che lo faceva lavorare in carcere, con una solidità, una fermezza e una capacità di accompagnamento che ha consentito a questo ragazzo una svolta. Tutto questo per dire che nel carcere non c'è un approccio che non possa essere che sinergicamente attento a tutti coloro che in quel luogo, con ruoli e scopi diversi, convivono di fatto ogni giorno. La questione della salute che è stata posta all'attenzione - i contagi sono veramente tantissimi in questo momento - ne è la conferma. Non si può curare soltanto il detenuto o soltanto il poliziotto: è evidente che tutto questo deve essere portato avanti in maniera unitaria. L'attenzione alla Polizia penitenziaria in questi tempi si è è manifestata con quella che da tutti è stata ritenuta la prima urgenza, quella delle nuove assunzioni.

migliaia le nuove unità che stanno per entrare in servizio o che saranno assunte con i nuovi concorsi appena sbloccati. Il 23

come non accadeva davvero da molto tempo. Non è accettabile un approccio al carcere che contrapponga detenuti e personale che lavora con loro. Insieme bisogna far progredire questo importante aspetto della nostra vita repubblicana verso l'unico obiettivo, che è quello indicato dalla Costituzione. Quanto alle osservazioni

soprattutto per i giovani detenuti, per i quali si è prevista la necessità di predisporre degli spazi dentro gli istituti minorili, aree attrezzate per riprodurre un ambiente il più possibile simile a quello familiare. Un altro aspetto a mio parere importante e a cui tengo moltissimo

nei luoghi geograficamente più vicini a dove ci sono gli affetti è un contributo importantissimo per poter alimentare quei rapporti che sono di sostegno al cammino di chi sta cercando di fare un percorso di rieducazione. Ancora molti altri interventi hanno toccato la questione del carcere. Al senatore Mirabelli vorrei soltanto replicare che c'è un incremento esponenziale del numero dei soggetti messi alla prova: 24.378 al 31 dicembre, mentre nel 2015 erano 6.557. anche un incremento continuo di posti disponibili per i lavori di pubblica utilità per le moltissime convenzioni che stiamo stipulando con diversi soggetti pubblici e privati. Uno degli ultimi che ho firmato è stata un'importante convenzione con il Ministero dei beni culturali, con il quale abbiamo previsto la possibilità di destinare a lavori di pubblica utilità le persone che devono scontare la loro pena o la loro messa alla prova in tutte le strutture dei beni culturali, musei o archivi, magari in opere di digitalizzazione. Ovviamente queste soluzioni danno un gran sollievo alle nostre amministrazioni, perché laddove c'è una carenza di risorse questa è anche una possibilità per portare a termine dei progetti altrimenti difficili,

di separazione o che riguardano la famiglia emergono elementi di contesto e il problema lo segnalavo solo per dire che ci devono essere dei raccordi tra le autorità procedenti. Il tema della violenza sulle donne è stato sottolineato dalla senatrice Cirinnà e dalla senatrice Rauti e sappiamo bene che è un'emergenza che veramente non tende a declinare e ci toglie il sonno, tanto diventa importante e grave.

Esso vuole affiancarsi al Codice rosso, che pure era una normativa già molto significativa per il nostro Paese, per completare un aspetto: prevenire prevenire tempestivamente i casi di violenza e di femminicidio. Non possiamo soltanto avere misure repressive e punitive. Quelle azioni violente vanno fermate. Da qui, come è stato illustrato della senatrice Rauti, l'uso del braccialetto elettronico, ma anche il maggiore uso del fermo, che normalmente si utilizza per altri scopi, solo dove c'è il pericolo di fuga, l'arresto obbligatorio e il necessario raccordo con le altre norme del processo penale; ma stiamo anche studiando una

è alla bollinatura della Ragioneria dello Stato, che ovviamente solleciterò perché possa arrivare al più presto. Posso immaginare che le date abbiano coinciso con il grande impegno sul bilancio, ma adesso è ora di sbloccare questo importante disegno di legge per consentire al Parlamento di portarlo a termine. Foggia è un caso gravissimo, non solo per le nove bombe di questi giorni. È da diversi anni che Foggia è al centro delle preoccupazioni di tutti, per il numero e per la barbarie di quanto avviene in quella terra.

parli, che la popolazione non abbia paura di guardare in faccia quello che c'è. Ho incontrato anche le due vedove Luciani, le vedove della strage di San Marco in Lamis, e gli imprenditori soggetti al *racket*. Sul punto specifico sottolineato, è oggetto di lavoro e devo dire che è stata una sollecitazione del sottosegretario Macina, nelle scorse settimane, quella di provare a individuare dei locali a Foggia, affinché quel *pool* di Bari che sta lavorando al caso (e che rimane sotto la Corte di appello di Bari, nel senso che non viene creato un nuovo ufficio giudiziario) possa essere localmente presente proprio lì.

una riorganizzazione della geografia giudiziaria per quella specifica situazione, ma di fornire dei locali fisici per marcare la presenza dello Stato e della giustizia in una terra che, in questo momento, è quella dove avvengono i fatti più efferati e clamorosi. Questo mi collega, però, ad altri interventi, della senatrice Gaudiano ma anche di altri, che mi hanno scritto da varie parti, ai fini di una riflessione sulla geografia giudiziaria. Un intervento organico, lo sappiamo, è stato fatto dieci anni fa. In questo momento stanno arrivando, dopo un po' di anni di sperimentazione, segnalazioni di vari luoghi dove quel disegno di razionalizzazione ha manifestato delle criticità e io sono favorevole a riprenderlo in mano come disegno organico. Ovviamente, sappiamo bene che nei

che è una componente non secondaria del rallentamento dei tempi della giustizia. In questa visione non sarei tanto favorevole a interventi scoordinati su singole situazioni, perché si rischia di creare maggiori irrazionalità a catena, ma una revisione può essere oggetto, a tempo debito, di una riflessione comune. ordinamento giudiziario e *referendum*, senatrice Bonino, l'ho detto dall'inizio: due percorsi legittimi, paralleli, hanno poche aree di sovrapposizione e bisognerà in quel caso vedere se il legislatore soddisfa le richieste dei *referendum* o meno; ci sono tutte quelle tecniche che ben conosciamo e il nostro impianto costituzionale queste forme di dialogo tra il lavoro in Parlamento, la democrazia rappresentativa e quella del *referendum.* Non è la prima volta che accade, ma su questo fronte ci sono anche tematiche distantissime che non sono oggetto della proposta dell'ordinamento giudiziario. credo nella sinergia delle due forme di intervento e di possibili riforme, quindi ben vengano entrambe in modo tale che entrambe siano portate avanti parallelamente. Spendo una parola su Chicco Forti (non so più che me l'aveva ricordato); era segnato nella relazione, non l'ho riportato qui perché ero già intervenuta varie volte nel dibattito pubblico su questo tema. Sono andata negli Stati Uniti a incontrare l'*attorney general*, il mio omologo a livello federale degli Stati Uniti, per dare di persona tutte le spiegazioni necessarie che loro chiedevano su cosa significhi applicare la Convenzione di Strasburgo in questo trasferimento di detenuti. Durante l'incontro c'è stato modo davvero di spiegare e chiarire ogni dubbio che potesse emergere. A questo punto siamo in attesa di una loro risposta, tenendo conto che questo tipo di decisioni negli Stati Uniti è complicato dalla struttura federale, perché deve esserci un assenso sia del governatore della Florida, che è il luogo dove è detenuto Chicco Forti, sia del Department of justice a livello federale, con il quale ho parlato. Con il governatore della Florida c'è una corrispondenza in atto e sto aspettando una risposta a una lettera che gli avevo scritto qualche mese fa. Non ci siamo dimenticati, è una persona che viene seguita, avevo anche parlato con la madre dopo questo viaggio; siamo in attesa di una loro risposta. Mi fermo qui. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma davvero non voglio approfittare della vostra pazienza. Qualcuno - se non erro la senatrice Modena - ha detto che è stato un impegno collettivo e il PNRR sarà ancora un impegno collettivo. Lo è. Siamo arrivati fino a qui attraverso percorsi che non era scontato ci portassero fin qui; è stato un anno in cui abbiamo riprovato a parlare insieme di giustizia. Credo che questo sia un risultato da non sottovalutare, possiamo parlarne, possiamo arrivare a dei testi; qualcuno ha sottolineato che non sono sufficienti, che c'è ancora tanta strada da fare: sono io la prima a esserne consapevole,

senatori, molti impegni rivolti al Governo corrispondono a linee di intervento già perseguite e per le quali sono già state adottate iniziative di riforme normative o attività istruttorie preliminari. Ne cito qualcuna perché si tratta di una risoluzione molto articolata: per esempio, l'attuazione del principio del giusto processo penale; nel civile, la decisione di tempi ragionevoli e abbattimento dell'arretrato. La riforma tributaria, come ho già annunciato, è una delle *milestone* del PNRR; c'è già una Commissione interministeriale che ha lavorato e dovremmo iniziare a considerarla dopo l'ordinamento giudiziario. Vi è poi il superamento di carenze dell'organico del personale, l'innovazione tecnologica e digitale: su questi e altri punti c'è una strada già già in parte percorsa insieme e che è ancora possibile percorrere, ma ci sono anche alcuni impegni che non posso condividere. Ne cito uno soltanto che è contrario alle linee di riforma adottate e sulle quali si sta lavorando:

il parere è contrario. Vi è poi la proposta di risoluzione n. 3, presentata dai senatori Gaudiano, Pillon, Mirabelli, Calienda, Cucca, Grasso e Unterberger, in cui, prendendo atto di quanto esposto e considerati gli impegni assunti dal Ministro guardasigilli, viene approvata la Relazione: su questa esprimiamo un parere favorevole.

di quello che nella Relazione è stato celebrato con un momento particolarmente alto: mi riferisco alla riforma della magistratura onoraria, che poi di fatto riforma non è, che non sta cogliendo nessuno degli aspetti che avrebbe dovuto cogliere nella realtà.

di un emendamento di tale portata nella legge di bilancio - perché avrebbe dovuto servire a bloccare la procedura di infrazione che era in corso in Europa. Lungi dall'ottenere quel risultato, la magistratura onoraria ha presentato un nuovo ricorso e, a sostegno della precedente procedura d'infrazione, ha mandato un altro documento nei giorni scorsi, che ovviamente è a conoscenza di tutti, nel quale si chiede un'ulteriore istruttoria da parte dell'Europa e quindi la prosecuzione della procedura d'infrazione aperta. Voglio ricordare anche che la magistratura onoraria ha proclamato uno sciopero, proprio contro quel tentativo di riforma, che partirà il 29 gennaio. È evidente che non è quello il metodo; il metodo avrebbe dovuto essere quello del confronto, il famoso emendamento sarebbe potuto arrivare in Commissione e probabilmente avremmo tirato fuori un provvedimento più efficace e completo.

di problemi. Mi riferisco, per esempio, al fatto della stabilizzazione che è soltanto apparente, all'introduzione di criteri per le retribuzioni che creano una disparità di trattamento perché ci sono quelli che possono svolgere un secondo lavoro, anche se non si sa bene quando lo dovrebbero svolgere considerato come vengono sfruttati i magistrati.

e a mettere mano davvero alla materia in maniera esaustiva e fattiva, perché solo in quel modo potremo dare una risposta a quelle persone, qualcuno addirittura da più trenta anni, bene o male vittime di una patologia del sistema. Avevano avuto infatti la possibilità di lavorare e lo hanno fatto. Chi parla è uno che da trenta anni osteggia la magistratura onoraria pensando che i magistrati debbano essere vincitori di concorso.

dell'assistenza contributiva e previdenziale. Questo è l'aspetto migliore del provvedimento, però ci si ferma lì e non si affronta il futuro. Questo aspetto ovviamente mi spaventa molto. esprimo grande apprezzamento sul processo di modernizzazione. Sappiamo perfettamente che i tempi della giustizia si ridurranno quando avremo la possibilità di attuare quel processo di digitalizzazione

credo che potrà essere uno degli elementi risolutivi. Ritengo che quello sia davvero un altro degli elementi su cui lavorare molto perché bene dice lei quando afferma che i tempi devono essere accorciati e in quel modo sicuramente si accorceranno moltissimo. Non mi voglio soffermare sulla riforma del civile e del penale, come ho già detto in precedenza. Deve andare a regime,

il tema in questione, come ripeto ormai da tempo perché è da anni che se ne parla e finalmente adesso ci si è avviati verso un percorso risolutivo, però dobbiamo metterci in testa che il tribunale della famiglia necessita di personale altamente specializzato.

un'attenzione particolare. Se vogliamo ottenere il risultato che auspichiamo, dobbiamo necessariamente mettere mano al personale amministrativo, ma ciò vale soprattutto per i giudici, che devono avere una formazione specifica per quel tipo di materia.

L'auspicio è che nell'adozione dei decreti attuativi, che dovranno essere portati all'attenzione per i prescritti pareri anche della Camera, si cerchi di superare il momento di stallo verificatosi sul tema della magistratura onoraria e il rapporto di collaborazione sia più fattivo di quanto sia stato fin qui. qui. È davvero necessario, infatti, che il parere del Parlamento venga tenuto nella dovuta considerazione, altrimenti siamo qui semplicemente per votare le fiducie e non per dare invece l'apporto che saremmo tenuti a dare. Mi è piaciuto molto anche quando lei ha detto che questa maggioranza è assai composita e che ha sicuramente una visione e idee differenti rispetto a molti temi delicatissimi della giustizia. Abbiamo passato la prima parte di questa legislatura ad assistere all'affermazione di un'idea più populista e demagogica (poi fortunatamente abbiamo superato questo tema), diretta più che altro a dare risposte al malcontento della gente. La giustizia non è questa; la giustizia deve essere fondata sull'applicazione dei principi costituzionali e in questo senso noi confidiamo molto nella sua persona. Lo ripeto spesso: lei ha esordito, nel primo incontro, dicendo che il suo faro è la Costituzione. Mi auguro che questo faro non manchi mai e le assicuro che da parte di molti di noi, direi di tutti quanti noi, questa sarà la frase che terremo scolpita nella nostra mente. Però - ripeto - alcuni provvedimenti hanno ostacolato oggettivamente una riforma che era stata avviata nella scorsa legislatura. Mi riferisco ad esempio alla giustizia riparativa. Sono molto contento che lei vi abbia messo mano, perché il tema dell'ordinamento penitenziario e della giustizia riparativa era stato totalmente pretermesso in sede di decreti attuativi; nella riforma Orlando, invece, esso era adeguatamente affrontato e ora saremmo già arrivati a una giusta conclusione. Dovremo ovviamente incentivare l'accesso ai riti alternativi, perché dobbiamo metterci in testa, come ho detto nella prima parte del mio intervento, che il carcere non è la regola, ma dovrebbe essere sempre l'*extrema ratio*. Quindi i riti alternativi devono essere sicuramente incentivati. È soprattutto necessario mettere mano anche alla materia dell'ergastolo ostativo, cui ho visto che lei ha prestato molta attenzione e di questo la ringrazio. Sono certo che riusciremo a fare un buon percorso; d'altro canto, è già all'esame della Camera. Infine, una parola sola sul CSM. Credo che mai la magistratura abbia attraversato un periodo di difficoltà estrema come quello che sta attraversando adesso. Anche gli ultimi accadimenti della scorsa settimana, dei quali non intendo parlare, confermano la crisi estrema della magistratura, con tutti gli accadimenti che conosciamo, e soprattutto di quello che avrebbe dovuto essere l'organo di autogoverno. Pertanto, è indispensabile che in tempi brevissimi si arrivi a una soluzione, ma a questa si può arrivare soltanto

è evidente che noi di Italia Viva - Partito Socialista Italiano voteremo convintamente a favore della sua relazione,

giustizia in Italia è drammatica. Non lo è da oggi e non lo è certamente per sua responsabilità, ma l'inefficienza e i ritardi della giustizia, come tutti sappiamo (anche lei vi ha fatto un breve cenno), costano costano in termini economici. Si pensi solo che, se la durata della giustizia italiana fosse paragonabile alla media europea, si calcola che questo produrrebbe 130.000 posti di lavoro in più; e sappiamo quanto sarebbe importante per l'Italia avere occasioni di lavoro in più. Ma soprattutto ciò rappresenterebbe un volano importante per gli investimenti dall'estero, perché sappiamo che purtroppo il tema della giustizia è uno dei principali ostacoli agli agli investimenti dall'estero in Italia (anche a questo lei ha fatto cenno). Eppure la situazione è oggi drammatica, come lo era un anno fa, signor Ministro. Certamente, ci sono stati

Abbiamo addirittura una spesa per ingiusta detenzione che supera i 27 milioni di euro all'anno: mille persone ogni anno finiscono in carcere da innocenti in custodia cautelare. Un terzo dei detenuti è in attesa di giudizio. Ci lamentiamo giustamente del sovraffollamento nelle carceri, ma un detenuto su tre oggi in carcere Sono temi, signor Ministro, che lei deve affrontare con maggiore decisione. Capisco che la sua è una maggioranza talmente ampia da contenere tutto e il contrario di tutto e questo purtroppo comporta spesso e volentieri dei compromessi al ribasso. Le riforme di cui lei ha parlato nella sua relazione sono al ribasso, signor Ministro. Lei è una giurista e non può non rendersi conto che, per tenere insieme tutto e il contrario di tutto, alla fine si arriva a individuare soluzioni assolutamente inadeguate. Lei ha fatto un riferimento e io non mi voglio sottrarre.

che c'è solo in Italia: avete messo insieme un istituto sostanziale come la prescrizione, fino alla sentenza di primo grado, e poi, per non scontentare i 5 Stelle, vi siete inventati la prescrizione processuale.

di consentire al giudice di secondo o di terzo grado di concludere il processo nei tempi della prescrizione, perché in appello la prescrizione non c'è più: ci sarà semplicemente l'improcedibilità. Quindi, da un lato, allungherete i tempi del primo grado di giudizio e, dall'altro, incentiverete l'appello, perché tutti appelleranno, nella speranza di beneficiare, poi, della prescrizione processuale, cioè della improcedibilità. Ecco un esempio per cui il compromesso, per una sorta di eterogenesi dei fini, produce il risultato opposto a quello che voi a parole

di portare in quel processo tutte le questioni che coinvolgono quelle parti. Ciò comporta che voi guadagnate tre, quattro o cinque mesi in quel processo, ma costringerete spesso quelle stesse parti a un secondo, un terzo o un quarto processo, per risolvere tutte le vicende che hanno in essere tra di loro. Vede come a volte, purtroppo, non avere una maggioranza coesa che va tutta in una stessa direzione porta a risultati paradossali, come questi? Certamente nelle riforme che abbiamo fatto

Per quanto riguarda il penale, penso alla presunzione di innocenza: vivaddio, finalmente! Finalmente ci sono dei criteri, per il rinvio a giudizio, che fanno riferimento non alla giustificazione del processo, ma alla ragionevole previsione di condanna: meno male! purtroppo, la situazione della giustizia in Italia ha comportato e comporta un crollo di fiducia degli italiani nei confronti dell'amministrazione della giustizia, perché non c'è solo un tema economico, di cui ho già brevemente parlato, ma c'è anche un tema di sentimento di giustizia, che oggi viene regolarmente calpestato.

Riformate come si deve il CSM: questo sistema elettorale delle preferenze multiple, a peso decrescente, sarà il trionfo delle correnti

la degenerazione correntizia, che è emersa dagli scandali di cui tutti purtroppo parlano. Allora si deve intervenire, a monte o a valle, ma troviamo il sistema: ci vuole il sorteggio! Basta con le porte girevoli tra magistratura e politica e prendiamo finalmente il coraggio di arrivare alla separazione delle carriere! *(Applausi)*. Signora Ministro, c'è un privilegio medievale, indegno di uno Stato di diritto, per cui i giudici godono di assoluta immunità: mi riferisco alla responsabilità civile dei magistrati. Dovremmo parlare piuttosto di irresponsabilità, perché anche nel caso estremo in cui un magistrato arrivi a rispondere dei danni che ha provocato, con dolo o colpa grave, tutti gli italiani rispondano con il loro patrimonio dai danni che provocano, il magistrato risponde solo nel limite di sei mensilità del proprio stipendio. è forse una vergogna questa? Signor Ministro, come possono pensare gli italiani di essere tutelati, se chi li giudica è immune e gode di un privilegio medievale. Ci sarebbero ovviamente tante altre cose di cui parlare, come la magistratura onoraria, calpestata e umiliata,

per cui un magistrato onorario che presenta domanda di stabilizzazione - vergognosa, perché li parificate al personale amministrativo - nel momento in cui presenta la domanda,

un imprenditore privato, con un suo lavoratore, il giorno dopo si troverebbe sotto processo per estorsione

precisi della nostra proposta di risoluzione, che indicano quella che dovrebbe essere la strada non di questa forza politica, ma di uno Stato serio e moderno che capisce che la giustizia è fondamentale per l'economia ma anche per la democrazia, perché senza sentimento di giustizia non c'è democrazia. *(PD)*. Signora Presidente, signora Ministra, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, condividiamo i contenuti e gli impegni presenti nella relazione e oggi è il giorno di un primo bilancio di un anno davvero intenso e difficile. Molte cose sono state dette dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dai colleghi del mio Gruppo Cirinnà e Mirabelli, quindi mi soffermerò

a lavorare insieme, a condividere, a decidere. L'abbiamo vissuto però fortunatamente non come uno sfortunato obbligo, ma come doveva essere, ossia come una grande occasione, una grande responsabilità per alcune riforme attese che dovevano - come è stato - essere discusse a lungo, condivise e decise insieme, in uno spirito di unità repubblicana e di grande responsabilità. Credo che questo spirito debba continuare e che si debba continuare con le riforme. Naturalmente, la parola magica di questa fase e del PNRR, per quanto ci riguarda, è la questione dei tempi. Un grande storico e intellettuale ha dipinto il passaggio allo Stato moderno richiamando il passaggio dei tempi della Chiesa in senso millenaristico ai tempi del mercante: che cos'è lo Stato moderno e che cos'è poi la rivoluzione industriale che è segnata dai tempi del mercante. Certamente la questione dei tempi in un'economia moderna, una economia della digitalizzazione, è un tempo folgorante da questo punto di vista, ma i tempi della giustizia italiana erano e sono ancora troppo lenti. Giustamente siamo intervenuti all'insegna di questa emergenza, di questa urgenza strutturale. Tuttavia, siamo intervenuti sui tempi con un grande obiettivo e punto di riferimento, e cioè che i tempi della giustizia hanno a che vedere con la piena attuazione dello Stato di diritto e dell'accesso ai diritti, tema che quindi non riguarda solo la giustizia penale, ma soprattutto la giustizia civile, alla quale abbiamo molto spazio e molta attenzione, perché la negazione dell'accesso ai diritti e i tempi troppo lunghi sono una negazione di giustizia e uno stravolgimento dei principi dello Stato di diritto. diritto. Quando parliamo di presunzione di innocenza, sono molto orgogliosa che abbiamo votato all'unanimità un orientamento del Parlamento sull'attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza. Lo si è fatto dopo una discussione, certo, dopo un ampio confronto, ma sono ancora più orgogliosa che nella riforma del processo penale questo sia stato uno dei principi informatori e parte della questione dei tempi, della ragionevole durata del processo. Troppa centralità è data alla fase delle indagini preliminari, troppa attenzione mediatica, e questo ha di nuovo a che vedere con la presunzione di innocenza; troppa marginalizzazione del processo, che è il luogo pubblico del difendersi provando, del contraddittorio, dell'attuazione delle garanzie. Vorrei quindi ricordare che il fatto che abbiamo riscritto che non si chiede il rinvio a giudizio se non c'è una ragionevole previsione di condanna, è un punto importante nel nostro percorso di riforme. Poi certamente c'è tutta la questione delle risorse, della modernizzazione e della riorganizzazione, perché per troppo tempo in passato si è discusso molto di giustizia come strumento di lotta politica e mai di risorse ad essa dedicate.

l'affermazione della laicità del processo. Lasciamo agli storici di studiare i processi, di fare ricostruzioni e di consegnarci delle elaborazioni, ma certamente sappiamo e affermiamo che non si fa la storia con i processi, perché i processi devono accertare verità, fatti e responsabilità e non servono a scrivere la storia. A questo principio ci siamo informati nelle riforme che abbiamo attuato. Parlando poi di modernizzazione, molto la novità di un dipartimento dedicato alla transizione digitale e alla statistica, perché questo implica una forma completamente diversa di organizzazione e anche un continuo esercizio nell'adeguarsi alle novità, tenendo conto tuttavia delle garanzie che vanno riscritte, ripensate e sempre tutelate.

dai diversi schieramenti si affermi che non va bene stare in carcere prima di essere giudicati, se poi addirittura si scopre che non si era colpevoli. Molto bene, quindi, che il carcere diventi un'*extrema* *ratio* come principio Naturalmente non è solo questo. Lei si è molto soffermata su questi punti e noi ovviamente vogliamo insistere per un intervento complessivo e organico.

nevralgico che ha a che vedere con la cultura delle istituzioni, che necessariamente dobbiamo condividere, pur nella differenza di opzioni, di prospettazioni e di proposte. Mi riferisco alla riforma del CSM. Non è da oggi che noi del Partito Democratico la chiediamo e su questo lavoriamo e avanziamo proposte. Addirittura già nella passata legislatura, con il ministro Orlando e con il contributo del nostro Gruppo, abbiamo presentato proposte articolate; oggi le abbiamo Non abbiamo quindi di certo aspettato i recenti fatti di cronaca per avvertirne la necessità o per avanzare idee e soluzioni. Possiamo certamente dire che questi ultimi due anni sono stati tra i più difficili che la magistratura ha attraversato nel rapporto con i cittadini, nonostante il lavoro dell'attuale CSM in senso innovativo e con spirito di responsabilità. Degenerazioni del correntismo, potere per il potere, un eccesso di autoreferenzialità sono i nodi venuti al pettine e che dobbiamo contrastare per contribuire a ricucire - come lei ha detto - quell'essenziale fiducia dei cittadini verso la magistratura e verso la giustizia. Consapevoli quindi di questa importanza e di questa responsabilità, pensiamo che non basti ovviamente cambiare la legge elettorale. Non si parla, quindi, certamente, soltanto di legge elettorale, ma ci vogliono una serie di interventi sulla riorganizzazione del lavoro che pensiamo, fra l'altro, non possa fare a meno del pluralismo delle idee necessario per la rigenerazione etica che non può, ovviamente, appellarsi soltanto a una modifica legislativa. È necessario il pluralismo delle idee contro la cristallizzazione del potere per il potere. Non basteranno, quindi, delle leggi sulla riforma elettorale.

della funzione disciplinare da quella delle nomine; proponiamo - tema sempre più presente nel dibattito di queste ultime ore sulle decisioni che hanno interessato il Consiglio di Stato e il CSM - l'istituzione di un'Alta corte con i criteri medesimi che adoperiamo per la composizione della Corte costituzionale, che si pronunci per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari e sulle controversie che riguardano tutti gli altri provvedimenti amministrativi, qual è per esempio quello dell'individuazione delle dirigenze degli uffici, per tutte le

la direzione, quali sono i principi, i punti di riferimento per queste importanti riforme che mettono al centro il rapporto tra cittadino e istituzioni? Qual è la cultura istituzionale condivisa, pur nella differenza delle idee? Credo che non possa che essere quella dell'autonomia e indipendenza della magistratura, della separazione tra i poteri dello Stato come garanzia contro ogni forma di arbitrio, per la tutela di tutte le libertà del singolo cittadino, sapendo che oggi discutiamo di questo nel quadro di un mondo che cambia, dove si accentuano le disuguaglianze con le conseguenti tensioni sociali e in queste tensioni sociali avanzano idee di uno Stato che superi la concezione democratica e liberale di Stati autoritari. Per questo è importante avere un quadro istituzionale di riferimento condiviso nell'indipendenza e nel controllo reciproco tra i poteri dello Stato. Tecnologie importantissime, che che però rimettono in discussione spazi personalissimi e che ci sfidano nella tutela di questi spazi e di queste libertà. Abbiamo bisogno di Abbiamo bisogno di rafforzare questi principi e non di picconarli, sapendo quali sono le criticità e qual è la cultura della laicità dello Stato, di una concezione liberale. Sappiamo che non siamo al secondo tempo di una partita cominciata più di vent'anni fa e non conclusa: siamo all'alba di una nuova era, con le sfide e le responsabilità che questo comporta e con quell'unità di intenti e di responsabilità istituzionale di cui non possiamo fare a meno e alla quale siamo chiamati a rispondere.

Ministra Cartabia, ascoltando la sua relazione non ho potuto non notare il riferimento che ha fatto alla costruzione dell'aula *bunker* del maxiprocesso alla mafia. Ricordo alla perfezione quei lunghi mesi di lavoro, animati dalla responsabilità di offrire a Palermo l'opportunità di celebrare il più importante processo penale della storia del nostro Paese. All'epoca, come giudice *a latere*, fui impegnato proprio nella supervisione di quei lavori e ottenemmo il risultato che ci eravamo prefissati proprio grazie allo straordinario impegno delle istituzioni che mostrarono, come mai prima di allora, un impegno concreto per combattere la mafia. La costruzione dell'aula *bunker* fu il primo passo; poi seguirono altri provvedimenti, come i primi *computer*, all'epoca strumenti di avanguardia, e tutti gli strumenti delle più moderne tecnologie che potevano aiutare e rendere più celere quel processo. Il Parlamento addirittura approvò, a tempo di *record*, una legge che ci consentì di superare le forche caudine del codice di procedura, che avrebbe messo a serio rischio il percorso del maxiprocesso. Quella straordinaria vittoria della legalità sulla mafia maturò, dunque, nello sforzo collettivo, seppure ispirata da due fuoriclasse come Falcone e Borsellino. Ancora oggi, il maxiprocesso testimonia come visione strategica, impegno collettivo e risorse bene allocate producano risultati straordinari. Oggi, dopo trent'anni, abbiamo un'altra occasione incredibile offerta dalle risorse del PNRR che giungono dall'Europa. Ed è proprio la dimensione europea che dobbiamo tenere a mente quando pensiamo alla strada che abbiamo davanti. A questo proposito, ho molto apprezzato il suo riferimento alla procura europea. Avendo in passato lavorato e collaborato alla sua realizzazione, essendo assolutamente convinto della sua importanza, non posso che essere felice e congratularmi per questo traguardo. Ella, nella sua relazione, ha descritto una visione del percorso di riforma del sistema giustizia che mi sento di condividere nei suoi obiettivi ma che, a mio avviso, non ha ancora ottenuto - ma è comprensibile - i risultati sperati. Io ho votato le riforme, pur non considerandole all'altezza della svolta innovativa di cui ha un disperato bisogno il sistema giustizia, ma comprendo come le situazioni parlamentari e la politica del momento influenzino talvolta le soluzioni. Serve, però, di più: seve ora e serve subito. Io sono convinto che vi siano due temi all'ordine del giorno di assoluta importanza, da lei citati, ma che meritano un'immediata risposta. Il primo è la modifica dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Si è iniziato un percorso, con una relazione della Commissione antimafia votata all'unanimità. Ora un testo è in discussione alla Camera. Serve coraggio, per evitare di dare una clamorosa opportunità alle mafie di rialzare la testa; serve fermezza, perché la lotta alla mafia è attualissima. Basti pensare alle recentissime notizie che giungono dalla Puglia, da Foggia. Serve fedeltà al dettato costituzionale. Lei ne è garante e ciò ci rassicura. Fedeltà che vede nello Stato il soggetto che amministra giustizia e mai vendetta. Io ho fatto delle proposte. Ho depositato un testo di legge in Senato e non posso che augurarmi uno scatto di orgoglio da parte del Parlamento prima che la Consulta intervenga ancora. Io non voglio neanche immaginare che a maggio, quando celebreremo il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, non sia ancora approvata una buona legge. Significherebbe macchiare, con enorme umiliazione, la memoria di quegli uomini e di quelle donne e ricordarli sarebbe una manifestazione di ipocrisia e non il tributo e il rispetto che meritano. Mi auguro che lo stesso coraggio serve per riscrivere le norme sull'ergastolo ostativo venga trovato anche per un'altra cruciale sfida che ci attende: la riforma del CSM e dell'ordinamento giudiziario. È in gioco la credibilità della magistratura, la fonte primaria della fiducia nella giustizia da parte dei cittadini. La composizione del Consiglio, pur avendo al proprio interno una naturale e, secondo me, necessaria dialettica di posizioni, che corrispondono ai diversi orientamenti, deve assicurare la realizzazione concreta dei principi costituzionali. Bisogna arginare il correntismo, partendo da una revisione delle norme relative alla elezione e al funzionamento del CSM, puntando sulla trasparenza delle procedure elettive di funzionamento. Penso a un meccanismo che garantisca la partecipazione più ampia a prescindere dalla designazione di gruppi organizzati, che premi il merito, la conoscenza dei problemi, che valorizzi anche la prossimità tra rappresentanti e rappresentati. Penso, poi, che si debba attenuare sensibilmente la possibile contiguità dei consiglieri con esponenti della politica attiva, inserendo delle limitazioni alla eleggibilità e all'accesso a incarichi direttivi, una volta terminato il mandato. Questi spunti, come lei sa, Ministro, sono contenuti in un disegno di legge che anch'io ho depositato in Senato. Abbiamo bisogno di un CSM autorevole per poter ridare credibilità a tutta la magistratura che paga come intera categoria le colpe di pochi, ma purtroppo influenti e decisivi magistrati. Signora Ministra, lei ha giustamente relazionato il Parlamento sulla situazione delle carceri. Quello che emerge, e purtroppo non sorprende chi, come me, per ragioni di servizio, le carceri le ha frequentate per tanti anni, è un quadro drammatico, e lei lo ha disegnato: carenza di spazi, carenza di personale, carenza di prospettive, carenza di speranze per il pieno rispetto di quanto previsto dalla Costituzione. Non ultimo - mi consenta di dirlo - carenza di cibo. Le gare d'appalto vinte a 2,39 euro al giorno di vitto per detenuto non sono solo anomale, sono indegne. Per questo ho apprezzato la separazione che nei prossimi bandi di gara si auspica tra vitto che, come risaputo, è a spese dell'amministrazione, e sopravvitto, che invece è a spese del detenuto. Credo che questa sia la strada giusta per consentire anche nelle carceri un'alimentazione adeguata.

ma come legislatori non possiamo non tenere conto delle enormi difficoltà di chi negli istituti penitenziari sconta la sua pena, ma anche di chi vi lavora quotidianamente. Le maggiori risorse stanziate, grazie anche ai fondi europei, sono certamente un'ottima notizia, ma nel tempo che occorre per l'adeguamento delle strutture - lo comprendiamo - abbiamo anche il dovere di garantire oggi il pieno rispetto dei diritti dei detenuti e di coloro che lavorano dentro gli istituti penitenziari. Il suo accenno in replica alla complessa vicenda di Chico Forti mi rincuora, e condivido con lei la speranza che possa concludere l'esecuzione della pena detentiva in Italia. Credo che questo sia il tempo di ritrovare quell'unità di intenti che segnò i grandi successi conseguiti ai tempi del maxiprocesso: visione strategica, risorse ben allocate, sforzo collettivo. Signora Ministra, le risorse ci sono, ingenti come mai nella nostra storia recente; la visione strategica che lei ha prospettato merita di essere perseguita, a patto che si realizzi per davvero e completamente, non solo in parte. Quanto allo sforzo collettivo, credo che questa ampia maggioranza, pure attraversata da una dialettica inevitabile e forte, debba assumere su di sé la responsabilità di trovare un punto di incontro che sia quanto più alto e concreto possibile. Non è il tempo di compromessi al ribasso, non è il tempo di tirare a campare; è il tempo del coraggio. A nome di Liberi e Uguali-Ecosolidali, esprimo il voto favorevole alla risoluzione n. 3, che prende atto degli impegni assunti e dei risultati raggiunti da lei illustrati.

la collega Modena ha già spiegato perché ci troviamo in un altro mondo, un mondo più felice da quando lei è Ministro della giustizia.

esistono due modi di essere parlamentari: uno è quello del parlamentare che vuole l'approvazione della bandierina, di un qualsiasi emendamento, che crede che l'attività legislativa che svolge il Parlamento sia affermare il credo del proprio partito. poi un altro modo, quello di credere e dare un supporto tecnico, politico, scientifico a quelle idee che vengono proposte da chiunque, ma che siano effettivamente nell'interesse dei cittadini. Forza Italia appartiene a questa seconda categoria e a questo gruppo di parlamentari. È questa la ragione per cui abbiamo sostenuto la sua idea di modificare il processo civile che ha introdotto la riforma del diritto di famiglia e istituito il tribunale della famiglia, che, quando sono entrato in magistratura nel 1970, era ancora un sogno; era quello che Maria Eletta Martini aveva già detto alcuni anni prima. anni prima. Ci troviamo di fronte però a un provvedimento per cui noi avevamo soltanto indicato, come ulteriore necessità per la sua funzionalità, alcune riforme: era la riforma della sezione tributaria della Cassazione. Mi scusi, Ministro, ma solo gente incompetente può dirle che si tratta di una questione che riguarda la riforma tributaria: non c'entra nulla. La Corte di cassazione civile svolge la funzione tributaria e quindi l'organizzazione della Corte appartiene al processo civile e lo sa meglio di me. Allora, c'è un problema di fondo che noi dobbiamo rispettare. Che cosa significava il disegno di legge sulle Camere arbitrali dell'avvocatura che accompagnava il disegno di legge del processo civile che doveva essere votato insieme? Devo dare atto a lei e alla struttura ministeriale di aver chiesto di rinviarlo, perché avremmo dovuto farlo a settembre, non perché non perché è stato proposto da un gruppo di senatori, ma perché quel disegno di legge significa alleggerire il carico di lavoro che c'è sui giudici ordinari. È questa la logica per far funzionare il sistema. Analogamente, se noi non alleggeriamo la sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo l'aumento del numero dei giudici che sono presso quella sezione, non avremo un sistema civile che funziona.

che era giusto fare una legge *ad hoc* entro il 15 gennaio, a cui avremmo dato un apporto tutti insieme, Parlamento e Governo,

di avere un ordinamento che risponde alle esigenze dei cittadini. Finalmente è stato approvato nella riforma penale un sistema che porta al riconoscimento delle sentenze europee che non avevano efficacia nel nostro Paese. Finalmente viene introdotto un sistema. Certo, resta ancora l'amaro in bocca di fronte ad alcune sentenze della nostra Corte di cassazione dichiarate illegittime a distanza di otto mesi dalla stessa Corte di cassazione e che però hanno esecuzione.

che alla base del sistema penale, per renderlo effettivo, bisogna eliminare l'appello del pubblico ministero alle sentenze di proscioglimento. Lo ha scritto Lattanzi

Il collega Dal Mas presenterà un disegno di legge, che ho sottoscritto anch'io, con il quale offriremo una soluzione al problema, al fine di renderlo compatibile con la vecchia sentenza della Corte costituzionale.

ma le chiedo di fare una commissione, un giorno, una seduta in cui il Senato possa esprimere le proprie osservazioni rispetto agli emendamenti che saranno presentati.

non è che noi abbiamo difeso e voluto le correnti solo per la pluralità delle idee. Le correnti in magistratura hanno determinato l'elevazione culturale e professionale dell'intera magistratura che invece prima era soltanto una selezione di pochi e per il resto erano tutti i burocrati. È questa la realtà. Noi abbiamo avuto una magistratura che si è elevata e ha potuto svolgere i suoi compiti a partire dal terrorismo e da Tangentopoli. da Tangentopoli. Tutto questo è stato possibile perché vi era una magistratura e le correnti che credevano nei principi costituzionali. Ministro, in conclusione vorrei esprimere un concetto: perché dico che non c'è e nemmeno le sentenze o gli atti di incolpazione che stanno valutando le ultime vicende della magistratura prendono in considerazione la questione? Quando sento che al Consiglio superiore della magistratura qualcuno sostiene che occorre andare a realizzare una discontinuità nella gestione di una determinata procura o di un determinato tribunale,

Quindi occorrerà valutare i sistemi di valutazione dei magistrati e i sistemi di nomina degli uffici direttivi. E, mi scusi, abbandoni l'idea dei piccoli collegi, perché la fine del Consiglio superiore è venuta proprio con i collegi rispetto al collegio unico nazionale.

Signor Ministro, è l'ora più buia della giustizia; è inutile che ce lo nascondiamo. Signor Ministro, io credo veramente che lei sia un Ministro competente, che lei sia riuscita a mediare anche posizioni inconciliabili e che lei sappia ascoltare. Però adesso le chiediamo di dimostrare un'altra dote: la dote del coraggio, perché, di fronte al caos che regna, servono riforme incisive e veramente coraggiose. Si è molto discusso in questi anni del conflitto tra la magistratura e la politica. Ma adesso, secondo me, c'è un conflitto molto più preoccupante, perché adesso c'è un conflitto tra magistrati.

altissimi magistrati da parte del CSM (stiamo parlando del primo presidente della Cassazione) e abbiamo avuto l'annullamento da parte del Consiglio di Stato. Pare che domani ci sia la rinomina da parte del Consiglio superiore della magistratura e probabilmente dopo ci sarà il ricorso avverso la rinomina. Stiamo parlando del primo magistrato d'Italia. Io non lo so chi ha ragione. Ho cercato di documentarmi e ho letto il più possibile: nelle motivazioni del Consiglio di Stato c'è scritto che il CSM avrebbe fatto una motivazione irragionevole, perché c'è un altro magistrato in corsa che aveva più titoli, il CSM replica con questa decisione che probabilmente sarà assunta domani e ha fatto trapelare, attraverso i giornali, che il Consiglio di Stato avrebbe travalicato i suoi poteri. Attenzione: domani c'è il *plenum* con il Presidente della Repubblica, che dunque deve scegliere se schierarsi con il CSM o con il Consiglio di Stato. Signor Ministro, io non mi schiero, ma prendo atto e chiedo a lei, che è Ministro della giustizia: cosa pensa di tutto questo? Cosa pensa di questi conflitti? Ecco, noi vorremmo che lei prendesse atto che non è tempo per i piccoli ritocchi. Noi vorremmo che lei prendesse atto che adesso servono veramente delle riforme profonde e radicali. Vede, quella del CSM non è una casa che ha bisogno di una ristrutturazione o di una tinteggiatura; quella del CSM è una casa da demolire e da ricostruire. Signor Presidente, sarebbe inutile un ritocco, mi creda. Ha dato prova di fallimento l'attuale sistema di avanzamento di carriera, che è quasi automatico. Ho sentito qualcuno che ha parlato già del sistema elettorale. Bene, io credo che a questo punto sia necessario introdurre il sorteggio, individuando dei requisiti iniziali per essere candidati. Quando si parla di sorteggio - non so se voi lo notate improvvisamente moltissimi si arrabbiano. Qual è l'obiezione che si fa al sistema del sorteggio? È la seguente: con il sorteggio si premia il fortunato e non il meritevole. Mi scusi, signor Ministro, ma l'attuale sistema elettorale ha premiato i meritevoli? Se avesse premiato i meritevoli - le dico di più - io preferirei i fortunati. Il sorteggio ha sicuramente un vantaggio, che è quello che consente di recidere il cordone ombelicale con le correnti eliminare evidentemente la gratitudine nei confronti della corrente che mi ha portato, quella gratitudine che mina per sempre l'indipendenza dell'eletto. La giustizia vuole certezze, signor Ministro, e noi stiamo vivendo nel caos. Non so chi di voi ha fatto una ricerca a fonti aperte, ma lei saprà molto di più di me, perché io ho cercato solo su fonti aperte le parole che mi vengono in mente: caos magistratura. Ed è venuto fuori questo: prima le cronache si occupavano di persone indagate dai magistrati; oggi si occupano di magistrati indagati da altri magistrati. Abbiamo pochi magistrati, ma quelli che abbiamo sono estremamente occupati in indagini delicate sui colleghi. Alla procura di Brescia, tra loggia Ungheria, caso ENI ed altre vicende, ci sono circa undici pubblici ministeri sotto indagine. I magistrati di Salerno indagano sui colleghi di Catanzaro, ma a sua volta un pubblico ministero della procura di Salerno è indagato a Napoli. A Perugia si indaga su numerosi magistrati romani; in Puglia c'è stata una sorta di record da quello che ho visto: nel 2021 ogni Provincia ha potuto vantare un magistrato indagato o condannato; a Trento circa sei magistrati; intanto a Caltanissetta ci sono i processi per i magistrati di Palermo sulla questione cosiddetta antimafia. Signor Ministro, queste sono ricerche a fonti aperte che può fare chiunque; chissà lei quanto indagini conosce. Io ho sempre difeso i magistrati e continuo a difenderli; sto parlando di alcuni magistrati. Attenzione: è indispensabile rimettere mano a una sezione disciplinare del CSM che faccia veramente il proprio lavoro. La giustizia domestica è inaccettabile per come, per ora, è stata realizzata. Con lei abbiamo anche parlato una volta di accesso alla magistratura lei propone di abbreviare i tempi. Gliel'ho detto e glielo ripeto qui: sono terrorizzata dal fare andare un laureato a ricoprire quegli incarichi; voglio che ci sia una valutazione di equilibrio, di scrupolo, di requisiti morali.

studiando tutte queste cose, a volte mi sembra che in questo momento la giustizia stia vivendo un po' come la trama delle favole di Gianni Rodari al rovescio, in cui non si capisce chi ha ragione e chi ha torto: Cappuccetto rosso è cattivo, il lupo è buono, c'era una volta un povero lupacchiotto che portava alla nonna la cena in un fagotto. Quando chiama al mio studio un magistrato, non so se chiama per un mio cliente o se lui vuole essere un mio cliente. Questo perché c'è caos, e tale caos si riverbera sulla quotidianità. Prima ai giovani laureati per spiegare il diritto si davano i manuali. Forse sarà capitato anche a lei che qualche ragazzo le chieda: come funziona il CSM? Io mi vergogno

come si vota di solito? Di solito si fa una votazione per decidere chi va in un posto. Poi ho pensato: ma perché devo mentire? Allora gli ho dato la *chat* dove c'è scritto: «Decidi chi va e poi organizziamo il voto». È possibile che dobbiamo dare le *chat* di Palamara per spiegare veramente come vanno le cose? a nove minuti e quindi devo tagliare, ma non posso non dire che nelle aule di giustizia campeggia la scritta «La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano».

Il popolo italiano sa - questo lo possono dire tutti gli avvocati - che il proprio avvocato parte sempre svantaggiato, nella migliore delle ipotesi, perché il pubblico ministero ha un rapporto di colleganza e di consuetudine col giudice; nella peggiore perché ci sono legami correntizi e magari il giudice ambisce a un incarico, che può ottenere solo grazie all'appoggio della corrente dell'altro magistrato *(Applausi)*. Ecco perché gli avvocati

sosteniamo anche la separazione delle carriere. Per concludere, signor Ministro, badi che ci sono tantissimi magistrati che lavorano silenziosamente, giorno e notte magistrati che non hanno avuto un incarico, perché sono fuori dalle correnti. Se quei magistrati oggi cominciassero a pensare che vivere onestamente è inutile, sarebbe la morte della giustizia. Voteremo a favore, ma le chiediamo coraggio!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Ministra, il momento storico nel quale ci troviamo impone, se possibile in maniera ancora più energica rispetto al passato, un'attenzione massima nell'adempiere al mandato ricevuto dagli elettori. Il protrarsi della situazione pandemica ha caratterizzato inesorabilmente l'attività legislativa e, tra i vari ambiti di azione dello Stato, anche quello dell'amministrazione giudiziaria è risultato colpito dall'emergenza sanitaria. Il legislatore, tramite una serie di riforme varate dal 2020 ad oggi - lo ricordo anche a qualche collega, che è intervenuto: dal 2020 - ha posto un argine, volto ad agevolare il corretto funzionamento dell'amministrazione. L'anno che si è appena concluso ha visto operare un Governo Governo nato per far fronte a tale situazione, composto da una maggioranza che ricomprende quasi tutto l'arco costituzionale e, per questo motivo, è molto eterogenea. Temi divisivi, come quello della giustizia, sono però stati affrontati avendo come unico obiettivo quello di riuscire a garantire l'efficienza del sistema. Molto è stato fatto, signora Ministro e infatti le diamo atto della completezza della relazione, ma molto c'è ancora da fare. Come Gruppo MoVimento 5 Stelle siamo contenti del risultato raggiunto con l'approvazione della legge delega di riforma del processo civile. Nella Commissione giustizia del Senato - come è già stato ricordato si è lavorato con una buona sinergia tra le diverse sensibilità politiche e il Governo è comunque riuscito ad armonizzare il testo in maniera organica. Un'esplicita dimostrazione è stata la ridefinizione della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, laddove si è riusciti a contemperare le quasi contrapposte esigenze di celerità e di efficienza del processo con l'effettività del diritto di difesa delle parti. Quello della legge delega, però, rappresenta solo un primo passo verso l'obiettivo di ridurre il 40 per cento del contenzioso e, appunto, il tempo medio di durata dei procedimenti. Sarà infatti solo con i decreti legislativi che si vedrà se questo percorso verrà realizzato o no. Sono interiormente contenta dell'approvazione di un emendamento, a firma del mio Gruppo, che ha previsto una procedura rafforzata in sede consultiva da parte della Commissione giustizia. C'è infatti l'esigenza, che comunque è stata anche rappresentata dagli altri colleghi che mi hanno preceduto, che si creino sempre di più una collaborazione stretta e una sinergia tra i Gruppi e il Governo.

A valle di un programma di rafforzamento degli organici del comparto di giustizia, che è già iniziato dal 2018 con il Governo Conte a seguito del varo del PNRR, gli uffici giudiziari stanno finalmente ricevendo quella linfa vitale di risorse umane senza le quali non può esserci alcuna riforma per accelerare l'*iter* dei processi e, quindi, abbattere il contenzioso arretrato, che purtroppo grava sulla nostra amministrazione giudiziaria. Siamo inoltre d'accordo con lei, signora Ministra, per quanto concerne il pronto recepimento della direttiva sul *whistleblowing*. Siamo stati infatti i primi a porre il tema al al centro dell'agenda politica quando, appena entrati in Parlamento nel 2013, abbiamo presentato la nostra proposta, poi trasformata in legge, e siamo contenti che il tema venga nuovamente affrontato. In relazione poi al monito della Corte costituzionale relativamente alle previsioni dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento giudiziario, il MoVimento 5 Stelle non può esimersi dall'intervenire, avendo come unico obiettivo quello di contrastare la mafia e la criminalità organizzata in generale, sotto qualsiasi forma si manifesti. Importanti pronunce della Consulta, infatti, vertono anche sui temi della diffamazione e, al fine anche di evitare la carcerazione per i giornalisti in caso di diffamazione a mezzo stampa e per quanto riguarda anche il suicidio assistito, vorremmo che in questa legislatura portare a termine quel percorso capace di portare alla luce provvedimenti in questi ambiti così importanti. A proposito della criminalità organizzata è stato messo in evidenza in alcuni interventi - anche lei lo ha ribadito nella sua replica la gravità dell'emergenza che si sta verificando nel territorio foggiano, dove c'è stata l'esplosione di diverse bombe che hanno inferto dolorose ferite alla comunità e lasciato ovviamente sgomenta tutta l'Italia, e non solo il territorio foggiano. Siamo di fronte a uno spietato attacco allo Stato, come ne abbiamo visti tanti anche in altre Province italiane. La risposta delle istituzioni, quindi, non può che essere perentoria, anche attraverso l'impiego di ingenti risorse umane e logistiche.

Più in generale ormai è il caso di fare un bilancio su quella che è la revisione della dislocazione dei nostri tribunali, visto che il risultato purtroppo è pieno di ombre. Mi fa piacere dunque che lei, signora Ministra, nella sua replica oggi abbia dato conto del tema e abbia comunque Sono evidenti le criticità legate al discorso della geografia giudiziaria, in termini sia logistici che di presenza sul territorio,

Per quanto riguarda invece il contrasto alla violenza sulle donne, molto è stato fatto, ma la strada è ancora lunga. lunga. La cronaca nera, infatti, quotidianamente ci ricorda che - se da un lato - esistono norme per salvare delle vite - dall'altro - purtroppo i risultati raggiunti non possono soddisfare tutti noi. Le norme ovviamente devono essere costantemente aggiornate e troppo spesso non vengono attuate.

della violenza nei confronti delle donne, che speriamo sia al più presto assegnato a una delle Camere, affinché si ponga quale strumento normativo atto a veicolare tutte le proposte sul tema a completamento di quello che era già stato previsto dal Codice rosso. Per questo è molto importante che veda la luce questo tipo di provvedimento. Per quanto riguarda la riforma ovviamente è già stata ribadita da più parti l'importanza che questo processo vada avanti. Sappiamo che è incardinato alla Camera e quindi auspichiamo che - come da impegno già preso all'interno della relazione - l'*iter* possa concludersi nel più breve tempo possibile, per ridare vita a un'istituzione importantissima per la nostra democrazia. Infine, desidero ricordare a tutti noi le parole pronunciate oggi da Papa Francesco a proposito delle persone detenute nelle nostre carceri: «È giusto che chi ha sbagliato paghi per il proprio errore, ma è altrettanto giusto che chi ha sbagliato possa redimersi»; «Non possono esserci condanne senza finestre di speranza». È quindi un dovere dello Stato tenere sempre aperta la finestra di speranza. Il carcere deve essere non solo astrattamente, ma con tutta la concretezza possibile, un luogo di reintegrazione di elaborazione degli errori e delle regole che disciplinano la nostra convivenza. A tale proposito, riprendo anche l'appello del garante per i detenuti Mauro Palma, secondo cui bisogna implementare anche all'interno delle carceri l'attività teatrale proprio come forma di risocializzazione e riabilitazione per i detenuti. ha parlato della pandemia come di una sfida dalla quale possono scaturire serie opportunità e spinte per il cambiamento. Le disposizioni speciali che hanno disciplinato l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria si sono rivelate in molti casi efficaci per consentire una più rapida trattazione dei processi civili e penali nel rispetto delle garanzie procedimentali e, al contempo, delle norme sanitarie vigenti.

in cui la giustizia non ha ceduto il passo alla pandemia, e questo per noi è importantissimo. Per questo, signora Ministra, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla risoluzione di maggioranza n. 3, a prima firma della Lo stato della giustizia in questo Paese, ossia il caos e il marasma di funzioni giudiziarie utilizzate come lotta di potere tra le correnti del CSM, giudicate dal compianto giudice Imposimato metastasi della magistratura, è stato plasticamente rappresentato ieri all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione. Dopo che il Consiglio di Stato aveva azzerato la nomina più importante del CSM - delibera del 15 luglio con le nomine del primo presidente di Cassazione Pietro Curzio e del presidente aggiunto Margherita Cassano, come se nulla fosse, nonostante le promesse di comportamenti più virtuosi e trasparenti nella designazione delle cariche dopo il gravissimo scandalo Palamara, il CSM ha deciso che il presidente Curzio potesse restare al suo posto a inaugurare la Caporetto della giustizia ingiusta 2022, sempre più a misura di potentati; aggravata, signor Ministro, dalla sua riforma, vera e propria *via crucis* per ladri di polli e poveri cristi senza santi in paradiso. Con la sua relazione ella indica come aggredire i tempi della giustizia penale e ridurre la pressione sul sistema giudiziario: l'improcedibilità in caso di condotte riparatorie, in particolare il risarcimento del danno. Da quanto emerge, non si intendono aggredire i tempi della giustizia con l'introduzione di soluzioni strutturali alle criticità riscontrate, illustrate dalla nostra risoluzione. Si preferisce invece selezionare i processi meritevoli di essere esaminati dal giudice o indicare l'improcedibilità di un caso giudiziario, estinguendo il reato, di fatto in violazione del diritto fondamentale europeo confermato tra gli obiettivi dell'agenda 2030: ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale precostituito. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Signor Presidente, sono l'unico dell'opposizione a intervenire. Ha consentito a tutti trenta secondi in più. Quella lotta spietata di potere e di poltrone tra le correnti della magistratura per accaparrarsi le direzioni più ambite, con alcune schegge impazzite di operatori certi di avere protezione dai loro capi corrente per i loro errori, ha prodotto anche il caso di David Rossi, suicidato, con i magistrati che, invece di indagare sugli autori e gli artefici, hanno indagato la moglie e un giornalista che aveva raccontato i fatti. Lei, signor Ministro, ha citato un eroe della magistratura. Se mi permette, cito Gratteri: se fossero in vita Falcone e Borsellino, immagino che salterebbero dalla sedia leggendo il termine improcedibilità in questa riforma, perché vuol dire che il 50 per cento dei processi in appello, dove c'è stata una condanna in primo grado, non si può celebrare. Nell'elenco mancano i reati ambientali, la corruzione, la concussione, il peculato, i reati che stanno gomito a gomito con la politica e con i faccendieri. Immaginate un operaio che cade dal quarto piano; viene condannato il datore di lavoro: è ovvio che questo processo in appello non si farà mai e andrà in coda. Mi devono spiegare quando avranno ristoro la vedova e i figli, quando avranno giustizia, dice Gratteri. A questo dovrebbe rispondere...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

abbiamo stabilito interventi a staffetta in Aula - per chi potrà anche sui suoi *social* - per non abbassare l'attenzione su quanto sta accadendo alle donne in Afghanistan. La Commissione diritti umani monitora continuamente gli avvenimenti e, purtroppo, dall'insediamento del Governo talebano, cioè dal mese di agosto, ad oggi, le condizioni di vita delle donne, nonostante tutti i falsi proclami,

a questo Senato l'attenzione che la questione merita e dico anche agli altri colleghi, al di là di chi siede nella Commissione diritti umani,

il materializzarsi di una situazione al tempo stesso triste e deleteria, che incide in maniera negativa sulla salute dei cittadini. La decisione adottata dai vertici regionali comporta la sospensione temporanea di tutti i ricoveri programmati nelle strutture sanitarie pubbliche: un provvedimento che - possiamo dirlo - sta già provocando e provocherà danni incalcolabili per tutti i pazienti affetti da patologie no Covid, che - come ben sappiamo - purtroppo, non sono per nulla scomparse. Anzi, sembra quasi un eufemismo, ma la cruda realtà è questa: si è oramai alzata bandiera bianca con il blocco totale o quasi dei programmi di prevenzione, con il calo della giusta attenzione per le patologie invalidanti e progressive, la cui ritardata diagnosi e il mancato giusto approccio terapeutico comportano ripercussioni non prevedibili e spesso non recuperabili e dagli esiti estremamente negativi per tantissimi malati. Questa decisione - secondo me del tutto inopportuna - è stata adottata per cercare di scongiurare nella realtà il collasso del servizio sanitario regionale e per camuffare anni di errori nella programmazione e nella cattiva gestione della sanità campana. E allora via solo ai ricoveri con carattere di urgenza, non differibili e non procrastinabili; per tutti gli altri restano pochissime alternative per cercare di superare il fattore tempo: lunghe liste di attesa o rivolgersi a strutture private. A questa situazione, già di per sé difficile e drammatica, si aggiunge, ad aumentare l'incertezza e lo sconforto dei cittadini, che l'assistenza territoriale, la quale dovrebbe fare da filtro per gli ospedali per evitare il loro logico tracollo, è quasi completamente saltata. Tutto ciò accade mentre scorrono nei nostri occhi le immagini di decine di ambulanze fuori dai pronto soccorso e delle file di persone in attesa per ore per poter praticare un tampone Covid. Sembra che due anni trascorsi dall'inizio della pandemia non abbiano insegnato nulla o quasi. Come nulla o quasi si è fatto per recuperare i *gap* iniziali e le gravi carenze strutturali ed organizzative della nostra struttura sanitaria regionale. regionale. Signora Presidente, ancora una volta la resilienza dipenderà, come sempre, dallo spirito di sacrificio degli operatori sanitari e dei cittadini, a cui va sempre il nostro ringraziamento.